L'ordine del giorno della seduta odierna prevede la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Al fine di consentire alla Commissione bilancio di terminare l'esame del provvedimento, la seduta sarà sospesa fino alle ore 13. Si ricorda che nella giornata di domani e di venerdì mattina l'Aula del Senato ospiterà la riunione del G20 dei Parlamenti. La prossima settimana, a partire da martedì 12 ottobre, alle ore 16,30, saranno discussi i seguenti provvedimenti: decreto-legge sulla crisi d'impresa, fin dalla seduta di martedì 12 se concluso dalle Commissioni; ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri; disegno di legge recante l'intesa fra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra; legge europea 2019-2020 con le connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; decreto-legge sulle modalità operative per la consultazioni elettorali del 2021, ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati. Il calendario della settimana dal 19 al 21 ottobre prevede - oltre al seguito degli argomenti non conclusi - nella giornata di mercoledì 20, alle ore 9, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021. È stato altresì stabilito che l'ordinaria programmazione del *question time* riprenda a partire da giovedì 21 ottobre, alle ore 15.

una nuova finestra"). Comunico che, su richiesta del presidente Gasparri, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

normalmente è un documento di assestamento in continuità con il DEF, ma quest'anno il quadro registra un riferimento macroeconomico di gran lunga migliore rispetto a quello del DEF, soprattutto grazie alla rimozione delle restrizioni sociali, grazie a un comportamento collettivo che ha permesso all'Italia di essere tra i primi Stati in Europa per tasso di vaccinazione e anche grazie all'utilizzo del *green pass*, che ha permesso la quasi totale ripresa di tutte le attività. Certo, il quadro spinto dalla domanda interna e dal commercio internazionale presenta comunque dei rischi che l'Ufficio parlamentare di bilancio, che pure

Sappiamo che in Italia e in Europa il tasso di vaccinazione è particolarmente elevato, ma un quarto della popolazione mondiale non è stato ancora vaccinato; quindi, non si può complessivamente scongiurare il rischio di varianti, né il rischio di variabili esogene e, di conseguenza, anche sull'economia. Un ulteriore punto che ha destato l'attenzione dei previsori riguarda l'inflazione, l'aumento dei prezzi sulle materie prime e sui semilavorati e anche una carenza nell'offerta di manodopera che, la tendenza, non supporterà a sufficienza, se non riadattata, gli investimenti previsti nella prossima legge di bilancio e anche quelli del Piano nazionale di ripresa Sul lato dell'offerta, il distanziamento sociale ha fatto moltissimo; altrettanto ha fatto l'incremento dei consumi,

anche dalla tendenza a investire e ad avere ottima fiducia sul futuro delle imprese. Per quanto riguarda la Nota di aggiornamento, il quadro macroeconomico tendenziale presenta, di conseguenza, un aumento significativo del prodotto interno lordo di oltre un punto percentuale superiore alle previsioni del DEF, e oggi pari al 6 per cento. Il prodotto interno lordo assorbe nelle proprie previsioni gli investimenti e le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e si attesta a livelli - anche nella prospettiva 2024 - molto superiori rispetto al *trend* storico che, purtroppo, sappiamo per l'Italia essere stagnante. Per quanto riguarda il quadro programmatico, la manovra di finanza pubblica continuerà ad essere fortemente espansiva, sicuramente per tutto il 2022 e per il 2023, con un grosso supporto alle famiglie e alle imprese per far sì che la la crescita sia completamente recuperata e che ci sia un consolidamento della crescita anche successivamente al recupero della caduta (ricordiamo pari a quasi il 9 per cento del L'elevata crescita è stata supportata anche dagli investimenti pubblici e molto dagli investimenti privati e dai consumi delle famiglie. Nella NADEF sono quindi presentate previsioni di finanza pubblica da cui deriva un miglioramento anche dell'indebitamento netto, che in fase tendenziale si porterà all'1,2 per a fine orizzonte, cioè nel 2024. Qualche dato anche su temi specifici rilevanti quale quello della pressione fiscale. Sappiamo che è stata approvata ieri dal Governo la delega fiscale, che si propone di rivisitare in maniera sostanziale vari aspetti del diritto tributario nazionale. Nel 2021 la pressione fiscale scenderà di circa 0,9 punti percentuali per poi stabilizzarsi negli anni successivi e tornare a ridursi gradualmente. Ci auguriamo naturalmente che l'effetto della delega fiscale e dei decreti legislativi che verranno attuati risponda alle attese delle famiglie e anche delle imprese. Per quanto riguarda la spesa pensionistica - altro dato rilevante in rapporto al PIL - sappiamo che è previsto che scenderà per cento solo nel 2024, ma ricordiamo che la spesa pensionistica era inferiore a questo dato, e cioè del 15,2 per cento già nel 2018. Questo incremento

molto a livello mondiale, soprattutto i Paesi altamente sviluppati, e interessa anche l'Italia. Su questo vale la pena ricordare che le previsioni registrano sì un aumento dell'inflazione dell'1,2 per cento nei primi tre trimestri dell'anno, che nel quarto trimestre, quindi su base annuale, è previsto un incremento dell'inflazione all'1,5 per cento, ma ad oggi il Governo e i previsori non ipotizzano che tale dell'inflazione sia stabile, quindi non prevedono effetti negativi sull'economia, sulla finanza e sui consumi. Tornando agli interessi, al di là di quest'anno, essi si ridurranno fino a registrare in rapporto al PIL il livello del 2,5 per cento nel 2024. Siamo consapevoli che è un livello assolutamente vantaggioso, soprattutto per un Paese con uno *stock* di debito pubblico alto come quello che l'Italia registra anche a seguito della pandemia. Questo ovviamente deve far sì che l'indirizzo di politica sia fare tutto il necessario affinché i bassi interessi aiutino l'Italia a ricondurre l'indebitamento pubblico verso un obiettivo di medio termine, nell'orizzonte prestabilito dalla NADEF entro il 2030 e soprattutto oltre il 2030. Per quanto riguarda gli altri punti fondamentali della NADEF, signor Presidente, noi non presentiamo una relazione di richiesta di ulteriore scostamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 12 del 243, perché fortunatamente l'andamento dell'indebitamento netto è negativo e comunque in progressiva riduzione. Non solo; tale andamento dell'indebitamento netto ci permette di liberare risorse consistenti per oltre un punto percentuale (1,2 nell'anno corrente, 1,5 negli anni successivi) tali da supportare e finanziare le misure che il Governo intenderà adottare in legge di bilancio, alcune delle quali saranno anche riassunte nella relazione di maggioranza. Ne ricordo qualcuna per punti perché sono misure fondamentali che fanno parte di riforme strutturali che il nostro Paese attende: la riforma degli ammortizzatori sociali, il primo pezzo della riforma fiscale e la stabilizzazione dell'assegno unico per i figli per supportare la natalità del Paese (altro dato che, oltre all'aspetto sociale, ha una rilevanza economica fondamentale). Inoltre si continua a supportare l'evoluzione e la transizione di tutto il settore produttivo e imprenditoriale con gli investimenti 4.0 e i vari fondi di garanzia. Ricordiamo che le politiche e i saldi strutturali di finanza pubblica degli ultimi ventiquattro mesi sono dipesi dall'attivazione della clausola di salvaguardia generale a livello europeo che ha permesso ai bilanci dei singoli Stati di adottare politiche di emergenza a supporto di famiglie e imprese, ma la deviazione dell'obiettivo di medio termine ovviamente avrà un termine e quindi, come la Commissione europea ha recentemente confermato, le politiche espansive e l'applicazione della clausola di salvaguardia saranno in vigore per tutto il 2022 si sta ragionando sul 2023. Il Governo ha più volte espresso grande impegno rispetto all'obiettivo fondamentale in questo senso, cioè la rinegoziazione e la riscrittura del Patto di stabilità e crescita a livello europeo. Se è vero che le regole economico finanziarie europee sono assolutamente indispensabili, è vero anche che quelle che precedevano la *general escape clause* non possono assolutamente essere applicate in questa fase. Per quanto riguarda il debito pubblico, esso anche grazie all'aumento del denominatore, quindi all'aumento del PIL, si riduce molto rispetto alle attese del DEF, di oltre 6,3 punti percentuali,

complice un leggero aumento dell'indebitamento netto, al 143 sia chiaro che la strategia di consolidamento della finanza pubblica si baserà principalmente, nei prossimi anni, sulla crescita del PIL, stimolata dagli investimenti, dai consumi e dalle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altrettanto chiaro che, a partire dal 2024, la politica espansiva dovrà diventare neutra, per poi tramutarsi in una politica economica e di bilancio più prudente, che ci porti a ridurre il rapporto tra debito e PIL e a registrare avanzi primari. L'obiettivo, che è stato esplicitato, per la realizzazione di avanzi primari è un contenimento della spesa corrente e un aumento delle entrate, ad opera di una più oculata lotta all'evasione, guidata e delineata dalla delega fiscale,

Mi preme sottolineare quanto sia fondamentale la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui effetti sono assorbiti nell'andamento del PIL,

e di governo locale, delle amministrazioni territoriali, ma anche delle precondizioni sociali e politiche, una sorta di stabilità

Grazie rappresentante del Governo, oggi assistiamo ad un atto gravissimo, di cui tutte le istituzioni che rappresentiamo devono rendere conto ai cittadini italiani. Il pericolo che era stato scongiurato con il precedente Governo, ossia quello di collegare l'autonomia differenziata alla legge di bilancio, ritorna oggi con la NADEF. In questo modo non solo si limita la possibilità per i parlamentari di esercitare l'attività emendativa, ma addirittura si pensa di impedire in futuro agli italiani di poter ricorrere al *referendum* abrogativo. Cos'è questo, se non un furto di democrazia? Non faccio mistero di aver sempre contrastato fortemente l'autonomia differenziata, perché non può esserci vera autonomia dei territori, se non si parte da una condizione di uguaglianza, la quale, come è sotto gli occhi di tutti, è lontana dall'essersi realizzata. Il Nord e il Sud sono ancora separati da un abisso: a Bologna abbiamo i binari sotterranei per i treni ad alta velocità, che arrivano e partono ogni mezz'ora; a Matera invece c'è la stazione, ma non ci sono i treni. A parità di abitanti, ci sono 66 asili nido pubblici a Reggio Emilia e solo tre L'alta tecnologia, la chimica e il manifatturiero continuano ad essere dirottati al Nord, come testimoniano le ultime scelte del ministro Giorgetti. L'ambiente e la salute continuano ad essere avvelenati dalla cultura dei pesticidi, dei fanghi e degli allevamenti intensivi, che al Nord concentrano il 70 per cento della produzione. I giovani meridionali, invece, sono costretti ad emigrare, portando con sé il loro tesoro di competenze e saperi, perché al Sud è stato fatto il deserto intorno a loro. Tutti ripetono che adesso arriverà il PNRR, ma peccato che, anche con il PNRR, quel 70 che in base alle linee guida di Bruxelles sarebbe dovuto andare al Sud, è dimagrito fin quasi all'anoressia. Questa non è propriamente eguaglianza o equità e, se non ci sono queste condizioni, l'autonomia differenziata si tramuta inevitabilmente in una secessione camuffata: la secessione dei ricchi, una vera catastrofe per il Sud e per il Paese intero. Si vuole scalfire il principio di unità nazionale, sancito dalla Costituzione, e noi parlamentari non possiamo permetterlo. Se l'autonomia differenziata dovesse diventare realtà, Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna acquisirebbero alcune competenze, stravolgendo l'assetto e il funzionamento dello Stato e svuotandone le attribuzioni. In questo modo si ridimensionerebbe la capacità delle istituzioni centrali di organizzare e gestire le politiche pubbliche in ambiti fondamentali per la vita del Paese. Non solo. Il progetto di autonomia, così come pensato oggi, prevede una riallocazione delle risorse fiscali al Nord molto più corposa, che naturalmente andrebbe a scapito del Sud. L'efficienza, il benessere e l'uguaglianza dei diritti fondamentali non possono essere beni limitati e la risposta a problematiche comuni a tutto il Paese non può essere l'attribuzione di maggiore autonomia e maggiori risorse solo ad alcuni territori, lasciando indietro gli altri. Non si può rompere il vincolo di solidarietà statuale, né cancellare il principio perequativo. Non può essere messa in discussione l'unitarietà della contrattazione nazionale. Sanità, prestazioni sociali, istruzione e formazione, lavoro e tutela dell'ambiente devono essere garantiti in tutte le Regioni attraverso una legislazione nazionale e con adeguate risorse. Definiamo prima i livelli essenziali di prestazione (LEP). Durante la pandemia la competenza regionale in tema di sanità ha mostrato tutti i suoi limiti e la lezione da trarne è che essa dovrebbe tornare in capo allo Stato. Il criterio della spesa storica non è adatto a garantire uniformità dei diritti, come dimostra lo stato esistente dei servizi pubblici. In Italia le gravi disuguaglianze nella fruizione di servizi pubblici essenziali dimostrano che la garanzia dei diritti fondamentali è completamente assente, oppure è condizionata dal territorio di residenza, con picchi di vera drammaticità nelle Regioni del Meridione d'Italia. Non si può pertanto concedere maggiore autonomia ad alcune Regioni senza aver adottato prima una legislazione nazionale che definisca leggi quadro sui principi fondamentali e garantisca in tutti gli ambiti i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi fabbisogni *standard*. *standard*. Quello che si cerca di fare oggi è intollerabile. Si vuole far ingoiare a forza una legge collegandola alla manovra di bilancio per liberare il percorso dai fastidiosi ostacoli frapposti dalla democrazia. Forse qualcuno deve pagare dazio ed è costretto a concedere questa benedetta autonomia differenziata, o forse alcune Regioni del Nord non hanno proprio intenzione di mandar giù il fatto che si metta finalmente mano ai LEP e che al Sud arrivi solo qualche briciola. Se ha ancora un valore la funzione che mi onoro di svolgere in quest'Assemblea insieme a tutti voi colleghi, farò tutto il possibile perché questo colpo di mano venga scongiurato. motivo, insieme ad altri colleghi senatori presenteremo un emendamento alla risoluzione di maggioranza per stralciare il disegno di legge sull'autonomia differenziata dal collegato alla manovra di bilancio.

ha un effetto devastante sulle prospettive di crescita. E la crescita si ottiene quando ci sono ottimismo e libertà. La crescita va suscitata e sarà l'unica soluzione al miglioramento e all'aumento delle entrate, perché ogni euro euro di contributo genera sicuramente subito 50 centesimi di restituzione allo Stato sotto forma di tasse ed effetti benefici con il resto, secondo il principio del moltiplicatore.

che esito avranno. Io penso che sia ora di dire basta: ci si vaccina e basta. Tutto il resto è noia, come diceva Califano. di bilancio dice anche che la tenuta del *trend* di crescita va sostenuta attraverso gli investimenti. Ci sono quei famosi 106 miliardi di residui passivi in conto capitale, che sono nel bilancio dello Stato e che, se solo le norme fossero più semplici, probabilmente potrebbero entrare in gioco. Poi c'è il PNRR, che è di 208 miliardi; in cinque anni, dal 2022 al 2026, sono 42 miliardi di investimenti all'anno. Saremo capaci di eseguirlo e di generare un effetto benefico sulla crescita? Le condizioni dell'Europa non saranno troppo esose? Saremo in grado di impegnare le risorse entro il 31 dicembre 2023, avendo realizzato i progetti esecutivi? qualche dubbio, se non troviamo la via per sveltire, indirizzare e dare entusiasmo e ottimismo. Una cosa che non ho mai capito e che sottopongo al Sottosegretario, molto attento, è come sia possibile che il PNRR provochi un aumento del PIL soltanto dello 0,4 per cento nel 2021 e dello 0,9 nel 2022. Una mole di investimenti di questo tipo

in aumento del 2,9 nel 2021 e del 3,1 del 2022. A me pare decisamente poco rispetto agli anni precedenti, che già erano di fermo cantieri.

in questo momento, per una fase di rimbalzo e comunque per gli effetti generali dell'economia mondiale, presenta un aumento maggiore rispetto al 4,5 previsto nel DEF.

più i 200 del PNRR e lo sfondamento di fine anno: ciò avrà un impatto mostruoso, se non ci sarà l'inflazione. La BCE dice che nel 2021 l'inflazione

con la certezza del voto di oggi, e poi siano trasportate nella legge di bilancio, perché questo avrà effettivamente un grosso impatto psicologico e un effetto di crescita. Auspico queste cose, ragionando con la testa mia e con quella delle persone che conosco, secondo buon senso, equità e massima disponibilità, conscio di essere maggioranza. Grazie

tramite un amento di diverse percentuali ripartite nei vari anni, nel 2024 si arriverà a scongiurare l'effetto negativo della pandemia. Qualora lo scenario futuro si rivelasse il più positivo tra quelli prospettati, nel 2024 arriveremmo a superare pienamente l'effetto negativo negativo della pandemia. Un intento dichiarato in questo atto è che la politica di bilancio rimanga espansiva fino a quando non avremo superato la crisi e che dopo diventi restrittiva in maniera virtuosa, nel senso di essere finalizzata alla riduzione del debito pubblico. Un altro obiettivo dichiarato è conseguire *surplus* di bilancio adeguati al raggiungimento dell'obiettivo espresso poc'anzi, ovvero la riduzione del debito pubblico. Ciò potrebbe avvenire solo in presenza di un *surplus* di bilancio,

arrivare a un aumento del gettito per l'erario. Evidentemente condivido l'obiettivo di combattere l'evasione, perché in questo modo si

competitività per il sistema, perché, non falsato dalla concorrenza sleale di chi non paga le tasse, evidentemente genera per

Questo lo dice la teoria e anche i nostri avi saggiamente dicevano che il buon pastore tosa la pecora e non la scortica, perché in questo modo rimane viva, produttiva e in salute, mentre scorticandola si ottiene un risultato maggiore subito, ma poi non si ottiene più nulla. Questa teoria popolare fu poi elaborata in maniera più scientifica da Laffer, che nella sua curva dimostrò in maniera inequivocabile, a mio avviso, come un aumento del gettito, superato il livello impositivo ottimale di tasse, porta a una riduzione del gettito, arrivando paradossalmente a introito zero per l'erario nel caso di tasse al 100 per cento, perché nessuno lavorerebbe per pagare solo le tasse. Queste due teorie di saggezza popolare ed economiche hanno avuto anche applicazioni concrete, perché Ronald Reagan, appena eletto Presidente, nel 1982, in attuazione della politica economica di Laffer, ridusse le tasse, ottenendo non solo un *boom* economico per gli Stati Uniti, di cui abbiamo tutti conoscenza storica, ma anche contestualmente un aumento del gettito per l'erario, perché in dieci anni si passò dai circa 600 miliardi del 1982 ai 2.000 miliardi del 1990, più del triplo di gettito, diminuendo le tasse. Non bisogna andare tanto lontano nel tempo o nel luogo per trovare esempi simili, perché, rimanendo in Italia, basta vedere ciò che è successo quando è stata introdotta la cedolare secca. La Ragioneria dello Stato sosteneva che non potevamo permetterci quella manovra, perché avrebbe ridotto il gettito: invece, la conseguenza è stata che il gettito è aumentato, perché i contratti sono stati registrati tutti. Se volessimo indicare un esempio al contrario, non dovremmo far altro che pensare a quanto accaduto quando è stato introdotto il superbollo. Nel 2006, in pieno furore ideologico della sinistra, che doveva far piangere i ricchi - ricorderete il manifesto con la scritta: «Anche

Perciò, dimostrato che aumentare le tasse non porta maggior gettito, ma il contrario, la strada che indichiamo è appunto quella opposta: stesso risultato, ma strada opposta. Parliamo di una strada percorribile, che getta

ho auspicato un'inflazione controllata per ridurre il valore sostanziale del debito pubblico, ma quella attuale rischia di essere una crisi inflazionistica senza controllo. Questo è dunque il momento per creare basi solide

Il PIL farà registrare un aumento del 6 per cento rispetto all'anno precedente, con un incremento dell'1,5 rispetto alle previsioni. Le esportazioni aumentano del 3 cento; aumenta la domanda interna, che si è molto rafforzata, mentre il *deficit* - altro dato molto importante - si attesterà poco sopra il 9, a fronte di una previsione di circa l'11 per cento. La crescita del PIL è attesa anche negli anni a venire e si stima che rimarrà positiva fino al 2024, che è l'orizzonte al quale si arriva con questa Nota di aggiornamento, dimostrando un'attitudine a una crescita consistente che nel nostro Paese era sconosciuta da decenni, segno quindi che tutte le misure che erano state approntate e approvate con il Governo Conte II andavano esattamente nella direzione giusta. Tutti questi dati vedono sostanzialmente concordi sia il Governo, sia l'Ufficio parlamentare di bilancio, sia gli organismi indipendenti, per cui possiamo affermare con una ragionevole certezza che il nostro Paese sta venendo fuori dalla grave crisi in cui era finito a causa della pandemia. Registriamo con grande soddisfazione la proroga del superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023, come noi del MoVimento 5 Stelle avevamo richiesto a gran voce, ma come avevano richiesto le imprese edili, gli artigiani, le aziende manifatturiere e i professionisti del settore. I dati del 2021 sono eccezionali: sono stati aperti cantieri per oltre 7 miliardi; tante nuove imprese edili si sono costituite per far fronte alla domanda e in tal modo si sta rispondendo concretamente all'esigenza di transizione ecologica e di diminuzione del consumo di risorse, specie quelle fossili, e di produzione di gas climalteranti. Noi del MoVimento 5 Stelle, che abbiamo ideato, proposto e poi fatto approvare questa misura, crediamo debba essere vagliato un ulteriore allargamento del superbonus, sia per centrare gli obiettivi di neutralità climatica che ci siamo dati in Europa, sia per creare lavoro e sviluppo davvero sostenibili per l'ambiente, sia, ancora, per rendere le nostre abitazioni più sicure dal punto di vista antisismico e più efficienti da quello energetico, sia, infine, per migliorare i nostri conti economici in merito al PIL, al gettito tributario e previdenziale e all'IVA. La nostra proposta, che facciamo a tutto il Parlamento e al Paese, quella di procrastinare ancora, dopo il 31 dicembre 2023, la validità del superbonus. Si tratta di una misura che sta esplicando appieno i suoi effetti e i dati dimostrano che non è una spesa per il Paese, ma anzi è una misura in cui davvero ci guadagnano tutti: lo Stato, l'ambiente e i cittadini. Sul fronte tributario, invece, stamani in audizione ho rappresentato al ministro Franco la necessità e l'urgenza di valutare con grande attenzione la possibilità di intervenire sulla sospensione dell'invio delle cartelle esattoriali, che - lo ricordo - ha avuto termine il 31 agosto, mentre il termine per pagare le relative imposte o chiedere la rateizzazione scadeva il 30 settembre. Ci sono tantissimi tra aziende, artigiani e famiglie che non riescono a stare in queste tempistiche, in questi termini, ma che sono contribuenti fedeli e onesti (che, tra l'altro, sono la stragrande maggioranza), i quali vogliono assolutamente versare le loro imposte, ma chiedono una diluizione delle tasse del 2020, perché gli effetti della pandemia per moltissimi sono stati devastanti. Credo che il Paese debba essere ragionevole e consentire a questi contribuenti onesti di superare l'attuale fase di oggettiva difficoltà economica. All'uopo, credo che sarebbe utile anche la cosiddetta rottamazione *quater* delle cartelle, di cui si parla da un po', che preveda quindi l'azzeramento di sanzioni e interessi, ma l'integrale pagamento dell'imposta, e sia riferita agli anni fiscali 2018-2019-2020. In tal senso, nei mesi scorsi ho più volte presentato emendamenti ai vari provvedimenti emergenziali che abbiamo approvato in Parlamento, ma finora senza esito. Davvero faccio appello a tutte le forze politiche e al Governo di raccogliere il grido di dolore di chi è in difficoltà...

appello a tutte le forze politiche e al Governo di raccogliere il grido di dolore di chi è in difficoltà, vuole pagare le tasse fino all'ultimo euro, però si trova in un momento particolare. Devo però anche registrare e stigmatizzare che, nel corso delle audizioni (e sono sicuro che sarà ribadito negli interventi che seguiranno il mio), è stato fatto, da parte dei partiti del centrodestra, il solito attacco al reddito di cittadinanza. È un argomento di cui si è parlato moltissimo in questi mesi. Salvini ed esponenti importanti della destra e del centrodestra; Salvini per esempio ha detto che presenterà un emendamento per cassarlo; Renzi addirittura sta promuovendo un *referendum* abrogativo, che però per la verità ha registrato finora la raccolta di pochissime firme, segno che forse nel Paese questa battaglia non è per niente condivisa. Il ritornello che è stato ripetuto fino alla noia è che il reddito di cittadinanza - a loro dire - andrebbe a mafiosi, delinquenti e a gente che non ne avrebbe diritto. Tuttavia, i dati ufficiali, che sono gli unici di cui dovremmo tener conto, smentiscono clamorosamente queste che, dal nostro punto di vista, sono menzogne vigliacche, in quanto solo il 3 per cento dei beneficiari è risultato irregolare. Sarei felicissimo, se si registrassero tassi di frode così bassi anche per altri sussidi e sostegni che lo Stato eroga generosamente ai cittadini e alle imprese, ma di cui non si parla mai,

non si troverebbero lavoratori stagionali, specie nei settori del turismo, della ricettività e della ristorazione; anche in questo caso, però, i dati smentiscono clamorosamente le chiacchiere che si fanno in giro al bar o nei salotti televisivi. Infatti, i dati ufficiali

contratti: nei primi sei mesi del 2021, si è registrato esattamente un *record* delle assunzioni dei lavoratori stagionali, cioè esattamente il contrario di quanto si va propalando in tv e a volte, purtroppo, anche in questo Parlamento. in questo Parlamento. Dopo questi dati inoppugnabili rispetto alle argomentazioni utilizzate dai nemici del reddito cittadinanza e del MoVimento 5 Stelle (perché il vero obiettivo attaccarci e tentare di delegittimarci), la nuova argomentazione è che il reddito di cittadinanza sarebbe responsabile dell'esplosione del lavoro nero, come ho sentito in audizione sia ieri sia stamane. Non avendo un solo dato a supporto, ma solo per fare becera si ripete ossessivamente che il reddito è responsabile di questa esplosione. I dati citati sono tutti falsi, mentre ho riportato quelli ufficiali, provenienti dall'INPS. Riteniamo particolarmente grave che si faccia questa propaganda a discapito di gente fragile e di nostri connazionali in situazioni di difficoltà, che meritano tutto l'aiuto che la comunità e lo Stato possono e devono dare loro. Ci aspettiamo pertanto che questo ignobile teatrino abbia davvero termine al più presto possibile. In conclusione, noi del MoVimento 5 Stelle continueremo a impiegare tutte le nostre energie con l'unico obiettivo di assicurare agli italiani una vita e un avvenire migliori. Continueremo a occuparci con particolare attenzione di quelli che hanno più sofferto in questi anni: gli artigiani, le piccole e medie imprese, chi lavora e sgobba ogni giorno, le famiglie e i cittadini. *(Applausi)*.

Il 29 settembre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e non vi era traccia del provvedimento recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, che invece ora si trova in cima all'elenco e appare sul sito del Ministero dell'economia

Non si dimentichi infatti che l'autonomia differenziata attribuirebbe alle Regioni competenze esclusive su materie essenziali, che inciderebbero sulla stessa unità del nostro Paese - si parla di ambiente, di salute, di salute, di lavoro e di scuola - accentuando quindi gli squilibri già esistenti, a cui ha fatto riferimento il collega De Bonis, tra le zone ricche e quelle povere del Paese e tra cittadini più o meno svantaggiati. Tutto questo va in contrasto con gli articoli 2 in cui si parla di

è fortemente limitata dai Regolamenti di Camera e Senato la possibilità di emendare il testo in Aula, essendo collegato alla legge di bilancio, per cui c'è una procedura rafforzata, che va seguita. Analogamente, il collegamento alla manovra di bilancio potrebbe far temere, a norma dell'articolo 75, comma 2, della Costituzione, che i cittadini non possano nemmeno far ricorso eventualmente allo strumento del *referendum* abrogativo. modo, va detto subito che, al di là della collocazione formale del disegno di legge, questa normativa è sicuramente e sostanzialmente ordinamentale. Tuttavia, in tal modo, l'Esecutivo di fatto conculca le prerogative del Parlamento e dei singoli parlamentari - segnatamente, di coloro che non sono membri delle Commissioni di merito - poiché la loro facoltà di emendare il testo sarà estremamente ridotta, in ragione della speciale speciale procedura prevista per i collegati alla manovra di bilancio, e con il tentativo anche di annichilire la sovranità popolare. L'effetto dell'approvazione di questa autonomia differenziata non potrà che consistere in una ulteriore privatizzazione dei servizi essenziali, aprendo ancora di più la via ai privati nel settore della scuola, della salute pubblica e del lavoro, nonostante quanto si sia tristemente e tragicamente evidenziato durante la fase più acuta dell'epidemia di Covid; come accaduto anche nella scuola, come già previsto in realtà nelle bozze che vennero discusse nel 2018-2019, prima della caduta del governo Conte I.

Deve essere consentito ai cittadini di esprimersi e soprattutto di conoscere il contenuto e gli effetti di questi provvedimenti. È molto semplice; questi provvedimenti non porteranno che alla balcanizzazione del Paese, alla divisione, alla creazione di tante piccole Italia in competizione tra loro, in competizione tra loro, mentre lo Stato non avrà nessuna capacità e nessuna risorsa per stabilire misure compensative. Noi stiamo facendo esattamente il contrario di quanto va fatto; prima ancora di stabilire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), La funzione pubblica deve consistere nell'impegnarsi a costruire, mantenere e rendere efficaci e sostanziali i diritti fondamentali e le grandi reti di servizio pubblico a partire proprio da scuola, sanità e lavoro. La funzione pubblica deve rimediare alle diversità e alle lacerazioni che la diversa opportunità di accesso al diritto crea nel nostro Paese. certamente in questo modo che si può agire. La funzione pubblica non deve accentuare, come sta facendo, attraverso l'autonomia differenziata, queste diversità. Si deve respingere questo ennesimo tentativo di sopraffazione anche del Parlamento che si ripete da parte dei vari Esecutivi. Ciascun parlamentare, secondo me, ha il dovere oggi di non abdicare alle proprie prerogative, ai propri doveri e, anzi, deve difendere la sovranità popolare nel contempo sia nella forma rappresentativa, qui oggi, sia in quella diretta che si esprime tramite *referendum* abrogativo.

importanti. Tutto questo è stabilito nella Costituzione ben prima dell'autonomia differenziata, che ne deve tener conto. Tutto questo deve essere portato all'attenzione dei cittadini attraverso un dibattito pubblico. Bisogna che il cittadino sappia cosa stiamo facendo, cosa sta facendo il Governo di questa Repubblica. Bisogna che cittadino sia informato per poter poi assumere le proprie decisioni. *(Applausi)*.

facendo implodere non solo la maggioranza che lo sostiene, ma pure le regole istituzionali e costituzionali, come poi spiegherò. Quindi ci troviamo ad esercitare il nostro ruolo, in un'Aula sempre più vuota, con un Governo rappresentato dalla degnissima rappresentanza del signor Sottosegretario, che ringrazio, che si trova però in assoluta solitudine, e in Commissioni parlamentari, quali quelle che frequentiamo, di

che le istituzioni dovrebbero dare, in momenti così importanti e difficili per il nostro Paese. Dunque, quando si analizza la Nota di aggiornamento al DEF,

se è vero come è vero che i dati positivi del DEF - come la collega Conzatti ha esplicitamente chiarito - sono determinati dall'aumento del PIL,

nelle zone basse della classifica europea, fortunatamente sono state messe da parte e i risultati si vedono nel DEF e, soprattutto, nella NADEF. Questo è forse l'unico aspetto positivo che mi sento di ricordare. Mi sento anche di richiamare le parole scritte dall'ex ministro dell'economia e delle finanze del Governo giallo-verde,

quando erano Ministri o comunque membri del Governo, coloro che prima e dopo dicevano e dicono queste cose, non erano in grado di realizzarle. L'ex ministro Tria, che so essere una persona seria, potrebbe spiegarci perché,

Credo che la risposta sia davvero *in re ipsa* e non serva una mia più esplicita considerazione. Continuo sul tema, dicendo che i tempi parlamentari

tra di noi e con il nostro popolo. Poi votiamo e avanti! Le regole della democrazia sono continuamente infrante,

nel quale vi è il rischio di totalitarismo. Tutte le regole della Costituzione sono state violate negli ultimi mesi e vengono vieppiù violate.

stato un atto di responsabilità verso la crescita del nostro Paese, che non ha colore politico, ma richiede solo una visione economica volta a dare prospettive vere all'Italia e all'economia nazionale.

nella maggioranza. Mi pare che i colleghi Ministri della Lega non abbiano partecipato, con un sussulto di orgoglio (benvenuto da parte nostra), alla riunione del Consiglio dei ministri di ieri perché il presidente Salvini ha detto

esattamente quando lo siamo noi parlamentari. Tutto si sta decidendo nelle segrete stanze di uno o due Ministeri. Questa è la violazione della democrazia, cari colleghi. Di che riforma vogliamo allora parlare? Di una riforma di buone intenzioni?

Fratelli d'Italia - mi permetta - chiede a ciascuno di noi e a ciascuno di voi, al di là del colore politico (lo ribadisco), un sussulto di orgoglio. Il Parlamento non può essere ostaggio di nessuno; non siamo mai stati a favore dei regimi autoritari e siamo i primi che sostengono la democrazia e la libertà. Vogliamo tutti insieme che non si arrivi non al partito unico, ma addirittura al *leader* unico, a colui o a coloro che nelle segrete stanze decidono le sorti di questo Paese. Non è accettabile. Viva la libertà, viva Fratelli d'Italia e il nostro Paese.

la Nota di aggiornamento al DEF del 2021 prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico. Si parte quindi dai numeri del Documento di aprile 2021, che vediamo migliorati nelle nuove previsioni.

La crescita del PIL, superiore alle previsioni di aprile, fa incrementare tutti gli altri indicatori di finanza pubblica; almeno per un po' si tratta ancora di un rimbalzo tecnico rispetto alla caduta dell'8,9 per cento del PIL nel 2020. A partire dal 2024 vediamo che la crescita economica si assesta all'1,9 per cento: un buon livello e comunque superiore a prima della crisi. È evidente che le previsioni di questa NADEF puntano sul buon utilizzo degli investimenti e sul raggiungimento degli obiettivi di riforma, nonché sulla volontà e la necessità di continuare con una manovra espansiva per i prossimi anni. La ripresa prevista negli anni 2022-2024 è sostenuta inoltre da un forte aumento degli investimenti, sostenuto anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il miglioramento degli indicatori previsti nel DEF e aggiornati nella Nota è sicuramente dovuto alla ripresa delle attività economiche, anche se nei vari confronti con le parti economiche e sociali emergono criticità che il Governo deve affrontare, per evitare un rallentamento dell'offerta sulla domanda. Sicuramente la più importante è dovuta al rincaro delle materie prime e ai colli di bottiglia della logistica internazionale, che rappresentano un forte freno all'attività globale. Sappiamo bene che proprio il rincaro delle materie prime e delle materie energetiche (luce e gas) va a incidere sui costi di produzione, con una ricaduta sul consumatore finale (famiglie e imprese), facendo balzare l'inflazione nell'ultimo quadrimestre al 2,6 Le misure messe in campo dal Governo, annullando transitoriamente gli oneri generali di sistema in bolletta e potenziando il *bonus* sociale alle famiglie in difficoltà, hanno di fatto tamponato in parte il problema sull'effetto diretto; ma rimane l'effetto indiretto, dovuto all'aumento dei prezzi sui prodotti di consumo. Altro tema sollevato è la difficoltà a reperire forza lavoro in tutti i settori, soprattutto i più trainanti (settore dei servizi e settore edile). Ricordo che il tasso di disoccupazione rimane molto alto, con il 9,6 per cento rispetto al 2020, che si attestava al 9,3 per cento. È urgente quindi un nuovo piano per le politiche attive, che introduca la revisione del reddito di cittadinanza, per colmare il *gap* tra offerta e domanda di lavoro. Ricordo che il reddito di cittadinanza è stato disegnato e voluto con l'obiettivo di mitigare la povertà, ma soprattutto per accompagnare i disoccupati nel mondo del lavoro. allo stato attuale non sta realizzando questi obiettivi, se non in misura molto limitata. A giugno 2021 c'erano 1,15 milioni di beneficiari, su oltre 3 milioni totali che avevano sottoscritto il patto per il lavoro; ma a febbraio 2021 solo 152.673 avevano instaurato un rapporto di lavoro. L'Italia non può vivere di sussidi; l'Italia deve vivere di lavoro e le aziende, insieme ai lavoratori, devono poter produrre. *(Applausi)*. Occorre intervenire sul cuneo fiscale per le aziende e sulla semplificazione per alleggerire il carico di burocrazia che attualmente grava in termini di tempo e denaro per le imprese. I dati contenuti nella NADEF ci dicono quanto siano state importante le misure di contrasto alla pandemia che hanno permesso una buona ripresa delle attività economiche. Sappiamo bene che una recrudescenza della malattia porterebbe a un crollo dei dati contenuti nella NADEF: una settimana di *lockdown* costa lo 0,5 del PIL. A tal proposito, ci preoccupa la diminuzione della spesa sanitaria al 6,1 per cento nel 2024, a un livello più basso del 2015 (6,6 per cento), dopo il picco al 7,5 per cento per le spese per affrontare l'emergenza pandemica. Con la pandemia molte persone hanno rinviato e, addirittura, rinunciato alle cure e non possiamo permettere che ciò continui a discapito dei soggetti più fragili e svantaggiati. L'attenzione per le problematiche concrete e imminenti da parte del Governo serve a infondere fiducia nei cittadini e può essere la ricetta per invertire la tendenza dei risparmi che le famiglie hanno adottato in questo periodo di pandemia - ricordiamo che i risparmi degli italiani ammontano a 200 miliardi - trasformandoli in investimenti e introducendo liquidità nel sistema. nel sistema. Presidente, l'impegno della Lega per un'Italia che cresce e vuole tornare ad eccellere in Europa e nel mondo c'è. Cerchiamo di continuare a fare politiche espansive, cercando di evitare vessazioni e tassazioni per le imprese che potrebbero ridurre questo buon andamento delle previsioni della NADEF. *(Applausi)*.

i dati presentati nella Nota di aggiornamento al DEF ci dicono che il maxi-indebitamento italiano inizia a scendere con un anno di anticipo. Anche questo ci deve far riflettere sul fatto

importante. Sono tutte riforme di contesto del sistema Paese che rendono effettivamente competitiva l'Italia e che rendono fruibili quegli investimenti, sia nazionali che internazionali, di cui c'è grande bisogno,

della popolazione. Questi sono due elementi su cui deve esserci poi una coerenza sulle priorità che ci diamo. Quali sono le priorità che io vedo dentro gli assi portanti

per aumentare l'occupazione, per creare buona occupazione, per creare un'occupazione stabile, qualificata e aggiungo - e di questi tempi non è un'aggiunta casuale - sicura.

che il Governo Draghi abbia incontrato le organizzazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e dell'impresa, mettendo al centro proprio questo tema, perché un lavoro deve partire dal fatto che nessuno può andare a lavoro e non ritornare a casa. Questo è un elemento fondamentale che porta

ripresa anche dalla relatrice in Aula. Dobbiamo sapere che c'è un asse fondamentale, a fronte delle analisi che tutti abbiamo sempre fatto delle insufficienze, del rapporto tra crescita e fabbisogno di competenze. Dobbiamo investire tantissimo sulle politiche attive del lavoro: deve essere questo il nostro asse. Investire sulle politiche attive del lavoro vuol dire creare una connessione nuova e più solida con le politiche formative, che devono essere sistematizzate all'interno di questo percorso, partendo dagli investimenti

storicamente si fatica a fare - la crescita economica, gli investimenti delle imprese in capitale con il capitale umano, che oggi è il punto di connessione fondamentale. Sappiamo che su questo abbiamo un'arretratezza molto forte. Questa scelta implica come conseguenza, perché è un intreccio mettere al centro le politiche per il lavoro come politiche di sistema, politiche di sistema, la riforma degli ammortizzatori sociali. Anche su questo spendo due parole: riforma degli ammortizzatori sociali, che devono coprire tutte le diverse fattispecie e accompagnare la transizione dei diversi processi, che in fasi diverse le imprese e le filiere produttive ricoprono.

riduce la povertà e le diseguaglianze; aumenta la ricchezza prodotta per tutte e per tutti, oltre all'autonomia e alla libertà delle donne, e ovviamente, con gli investimenti nelle infrastrutture sociali, produce esattamente un'inversione della curva curva demografica. C'è bisogno però che tutto il Paese sia coinvolto in questo straordinario processo di cambiamento. Pertanto, io non amo usare la parola «patto» in astratto. Il patto di Ciampi, a suo tempo, aveva una finalità diversa; il dialogo sociale in Europa aveva una funzionalità diversa. Oggi stiamo parlando di un coinvolgimento democratico di tutte le istituzioni che hanno responsabilità istituzionali e sociali, sia a livello nazionale che a livello territoriale, perché questo è il grande cambiamento che si può solo governare insieme, ciascuno per le sue funzioni e responsabilità, ma è altrettanto importante. Diversamente, anziché anziché utilizzare al meglio questa straordinaria opportunità di risorse, rischieremmo soltanto di aumentare il divario e non affrontare il *gap* che questo Paese ha di fronte.

ed è un'importante iniezione di ottimismo per tutti quei soggetti che operano nella nostra economia. Senza ottimismo è difficile poter investire ed è difficile poter creare lavoro. Prima di entrare nel merito, vorrei soffermarmi su alcuni punti sfiorati in Aula da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. L'Europa è vero che è stata silente e sorda ai tanti richiami, è inutile nasconderci, però c'è qui dentro chi si è diviso tra coloro i quali chiedevano un'Europa più vicina, più forte e più unita, e chi chiedeva addirittura di uscire dall'euro e dall'Europa. Oggi sembra preistoria, ma fino a un anno e mezzo fa sentivamo questi discorsi in quest'Aula. Il clima dell'austerità, che purtroppo ha persistito e ha profondamente danneggiato coloro i quali credono in un'Europa più forte, a nostro modo di vedere, si è inclinato con la guida di Draghi alla BCE: è inutile nascondercelo. Draghi ha salvato l'euro e ha salvato l'Europa con il *quantitative easing*. Questi sono dati che sarebbe sbagliato trascurare. Certamente la pandemia - altrimenti sembra che viviamo una realtà diversa - ha accelerato questo processo,

per cui bisogna accettare quei parametri del 2,04 (col trucchetto 2,4), perché purtroppo o per fortuna viviamo in una comunità di regole ed è strano che proprio chi auspica il rispetto delle regole poi chieda delle deroghe. Mettiamoci a parti invertite:

si firma un trattato e si vuole essere credibili nello scacchiere interazionale lo si deve rispettare; poi si può combattere per modificarlo, per allargarne le maglie, ma di certo non si può non rispettarlo, anche perché i danni, se non lo si rispetta, non li paga il Presidente del Consiglio o il singolo senatore, ma un Paese di 60 milioni di abitanti.

che si poteva evitare), abbiamo espresso le nostre perplessità non sull'entità e su una sorta di reddito di inclusione, ma sulla modalità con cui questo si andava ad espletare, perché si fondava su due pilastri: il sostegno e l'assistenza e le politiche attive del lavoro. Quelle, amici miei, non ci

i 7.000 *navigator.* Chiunque di noi abbia la possibilità di farci un dialogo si rende conto che non combinano nulla, non perché siano dei nullafacenti o degli incapaci, ma perché non hanno gli strumenti per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. *(Applausi)*. È tutto lì, non è un atteggiamento pregiudiziale o ideologico, come qualcuno di voi vuol far pensare. cuba 7 miliardi di euro l'anno), per carità di Dio, è ottimo, è buono, ma non può essere sufficiente esclusivamente la contemplazione di un provvedimento che non funziona, così come tanti altri provvedimenti non hanno funzionato durante la pandemia - è inutile nascondercelo - e sono stati migliorati,

perché la sensazione che si ha è che le attività commerciali e le aziende continuino a chiudere; quindi, qualcosa in quel meccanismo dei grandi numeri non funziona; non so se sia l'incapacità di aggiornamento, di formazione, di reinventarsi, però qualcosa non funziona. La riforma fiscale è un tema delicatissimo, perché questo è un Paese che se non cancella l'ipocrisia del rendere conveniente dichiarare piuttosto che non dichiarare, non ci sarà una riforma fiscale adeguata.

una sola preoccupazione. L'elemento devastante è l'incremento del prezzo delle materie prime e dei costi dell'energia. Bisogna prestare attenzione perché un'inflazione troppo alta, con il rischio di una stagnazione, crea le condizioni crea le condizioni per una tempesta perfetta. Io sono convinto che il Governo stia adottando l'eventuale piano B, i due pilastri su cui si fonda sono maggiori investimenti e minore pressione fiscale, quindi due leve variabili, ma suggerirei un intervento corale dell'intera Unione europea per far fronte a questa minaccia. *(Applausi)*.

Infatti, dall'Ufficio parlamentare di bilancio ci dicono che il quadro macroeconomico del MEF è quantomeno lievemente ottimistico rispetto alle previsioni, e non solo per il rischio pandemico, ma anche per degli inasprimenti degli inasprimenti differenziati delle politiche economiche. Ciò significa che, finita la pandemia, finiranno le politiche espansive di Governi e banche centrali, e banche centrali, e il riassorbimento degli squilibri finanziari accumulati, ossia i debiti, in tempi che potrebbero essere troppo affrettati potrebbe portare a gravissimi sfasamenti nei cicli di ripresa dei Paesi. In Italia, lo *stock* di debito pubblico è elevatissimo e le tensioni finanziarie potrebbero velocemente interagire con la ripresa. Questi rischi dipendono molto dal nuovo sistema di regole di bilancio, sulla cui revisione occorre perciò concentrare la massima attenzione e cautela. Detto questo, quello che vogliamo sottolineare nel poco tempo che abbiamo a disposizione

di trasformazione della *green economy* e dell'economia circolare (la famosa *green generation*), su cui nella precedente formazione di Governo stavamo lavorando perché era il collegato ambientale alla legge di bilancio precedente. di legge in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva. Si tratta di iniziative legislative fondamentali per la transizione ecologica e per la tutela dei diritti dei lavoratori; temi prioritari e irrinunciabili per il raggiungimento degli obiettivi di equità e giustizia, sociale e ambientale, che ci raccomanda l'Europa. Eppure, si legge testualmente che, per effetto della mancata previsione nella NADEF 2021, questi cessano di essere disegni di legge collegati alla decisione di bilancio. È una cosa gravissima,

Soprattutto - così come hanno già detto i colleghi in precedenza - c'è una cosa che non dovrebbe esserci: ancora una volta, alcune Regioni tramano sottobanco - come abbiamo detto in un comunicato stampa a danno dell'unità della Repubblica. Il pericolo era già stato intravisto e superato con il precedente Governo, in particolare con il ministro Boccia, che aveva provato a collegare l'autonomia differenziata con la legge di bilancio. Oggi il Governo Draghi ci torna, dovendo probabilmente pagare dazio, e ripercorre lo stesso tentativo nella NADEF: interferisce e inserisce tra i ventuno collegati il decreto-legge "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione". È il primo disegno di legge nell'elenco, quasi a significare che la sua approvazione ha carattere prioritario. Eppure, è stato inserito in assenza di un dibattito pubblico; anzi, direi di più: in spregio delle considerazioni emerse dal dibattito pubblico che c'è stato durante la pandemia da Covid-19, che ha evidenziato i profondissimi limiti di efficienza e di coordinamento - ce lo ricordiamo tutti del decentramento delle funzioni con riguardo a valori fondamentali come la salute, l'ambiente, l'istruzione, il lavoro, valori tutelati dalla Costituzione. che, con le autonomie, renderebbero ancora più grave il divario esistente tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia; graverebbero enormemente anche sulla ripresa del Nord - questo lo dicono tutti gli osservatori economici e ulteriormente sulla violazione del principio di uguaglianza - già violato - di cui all'articolo 3 della Costituzione. Ha carattere prioritario non l'approvazione del disegno di legge in oggetto, ma la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali che aspettano da trent'anni. Abbiamo messo a punto un emendamento in tal senso, che presenteremo al più presto, per lo stralcio di questo collegato. Non è il momento di affrontare, con un Parlamento commissariato da una maggioranza bulgara, una delle questioni più scottanti per il Paese; un presupposto che nasce da una modifica del Titolo V valutata errata da più parti, che sarebbe ora di mettere al centro del dibattito

per sottolineare come, ancora una volta, i tempi siano troppo compressi. *(Applausi)*. Non è pensabile fare l'analisi della NADEF, che nelle altre occasioni

Come potrebbe essere diversamente con le misure e la potenza di fuoco messe in campo? La preoccupazione emersa durante le audizioni anche dagli

degli atti precisi, come lo è certamente - lo diciamo da anni in quest'Aula - il contrasto all'evasione fiscale. Bisognerà, poi, porre particolare attenzione all'aumento della spesa per gli investimenti,

di avere un livello di base che ci proietti in un futuro di maggiore benessere. Certamente sono molti i problemi, e ne tratterò solo alcuni.

perché devono poter rientrare quelle persone - le donne soprattutto - che sono state espulse a causa della pandemia; ma bisogna che ci sia anche una formazione particolarmente efficace di tutti i lavoratori. Se il nostro deve diventare un Paese con conoscenze digitali più diffuse; se il datore di lavoro - industriale, artigiano, pubblica amministrazione - richiede un livello maggiore di conoscenze, di abilità e di produttività, bisogna che queste siano sostenute da un livello di istruzione e formazione crescente. Quindi, dovremmo davvero concentrare le nostre forze, le nostre risorse e i nostri investimenti su questo

trovino incentivi che li portino a rientrare nel nostro Paese. Il clima di fiducia e di aspettative positive ora c'è:

Paese. Bisogna fare in modo che quei ragazzi che si sono formati in Italia o all'estero, ma che comunque ora sono all'estero, tornino e diano il loro contributo alla crescita di un Paese che si sta muovendo,

possano essere adeguati a ruoli migliori, comunque più performanti. Quindi, si alza il livello di tutti i lavoratori. E questo è ciò che dobbiamo fare per programmare

ma soprattutto il costo è enorme: 7 miliardi all'anno. Forse sarebbe meglio pensare all'educazione scolastica, ad aiutare le famiglie con ragazzi disabili

chi ha ricominciato a investire, a esportare, a produrre, a cercare anche sistemi più sostenibili per fare impresa. Occorre

2021 non può non tenere conto che la situazione economica e sanitaria è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Tutto ciò è innegabile ed è avvenuto con il concorso di diversi fattori che hanno influito più che positivamente sul percorso di ripresa globale del nostro Paese. Le misure di sostegno economico alle attività in crisi e il progredire della campagna vaccinale con il coinvolgimento della fascia di età adolescenziale e dei giovani hanno permesso di far fronte alla quarta ondata e alla diffusione della variante Delta, molto più contagiosa. L'obiettivo di vaccinare l'80 per cento della popolazione sopra i dodici anni sta per essere raggiunto. Nel programma del prossimo triennio 2022-2024 è previsto il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, come - ad esempio quelle relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e gli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici, misura quest'ultima voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle. Più in particolare grande valenza avranno le misure relative al nostro sistema sanitario, al suo funzionamento, al miglioramento dei servizi erogati sia in termini qualitativi che quantitativi, ai criteri direttivi per il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico; a una più attenta programmazione e a una più capillare rete organizzativa sul territorio con il conseguente potenziamento della medicina territoriale, vero spartiacque per ottenere un innalzamento dei servizi erogati e una riduzione dei carichi di lavoro delle strutture ospedaliere. Si tratta di un progetto ambizioso, alla cui realizzazione devono concorrere un'adeguata disponibilità di risorse economiche - messe queste ultime a disposizione dai fondi europei ricevuti con il PNRR e ottenuti dall'Europa grazie al Governo Conte II II - e il corretto coordinamento tra la cabina di regia centrale e le singole strutture regionali. Solo una più attiva e fattiva collaborazione tra Governo, Ministeri e Regioni, che tante volte è venuta meno durante la fase acuta della pandemia o si è scarsamente realizzata per veti incrociati o anche per scelte politiche periferiche diverse, consentirà di iniziare un percorso nuovo e di raggiungere obiettivi e risultati non altrimenti realizzabili. Non dobbiamo mai dimenticare le oltre 130.000 vittime della pandemia da Covid-19 in Italia, 4,5 milioni nel mondo, con oltre 225 milioni di contagi. La scelta dell'estensione dell'obbligo del permesso sanitario a tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati, a partire dal prossimo 15 ottobre, va secondo me nella giusta direzione di stimolare e incrementare la pratica vaccinale da un lato - anche delle fasce più reticenti e - dall'altro - soprattutto la necessità di una sempre più attenta e costante sorveglianza epidemiologica al fine di ridurre i contagi e la diffusione di eventuali varianti del virus per sconfiggere finalmente la pandemia. Saremo protetti quando tutti saranno protetti. A tal fine, anche l'avvio delle terze dosi di richiamo ai soggetti più fragili prima dell'inizio dell'inverno e una più estesa e diffusa campagna vaccinale per l'influenza stagionale consentiranno di abbattere i rischi di nuove ondate epidemiche, con sovraccarico delle strutture sanitarie ospedaliere. Tutto ciò ha un costo economico, ma l'iniziale incremento di spesa sanitaria per il 2020, a seguito delle misure introdotte per dare immediate risposte all'emergenza da Covid-19, nel 2021 sarà seguito da una prevista lieve discesa della stessa spesa sanitaria, per cento del PIL, fino a ritornare, per il 2024, al 6,1 per cento. Tutto ciò è legato sostanzialmente all'aumento generale del PIL. Nel prossimo biennio si prevedrà prevedrà un calo del 2,3 per cento della spesa sanitaria, per i minori oneri legati all'emergenza pandemica. Concludendo, signor Presidente, al di là delle cifre e dei numeri, pure importanti, ciò che interessa ai cittadini e quindi al Movimento 5 Stelle è è constatare e toccare con mano ogni giorno che le risorse siano investite e impegnate nel modo migliore, in termini sia di servizi, sia di attenzione alle criticità, alle fragilità e alle disabilità.

la discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza credo rappresenti, in questo contesto, un decisivo momento di confronto politico. Se non cogliamo questo aspetto, rischiamo di procedere con alcuni fraintendimenti, che potrebbero amplificarsi e diventare disgreganti nell'interpretazione del percorso che il nostro Paese ha intrapreso, attraverso il Governo Draghi. Draghi. Vedete colleghi, quello che abbiamo iniziato è un percorso che ha degli obiettivi chiari, sui quali non mi soffermo, perché credo che ne abbiamo discusso molto. Essi sono scritti nel contratto che abbiamo fatto con l'Unione europea, che si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. In base a quel contratto stiamo ricevendo le risorse del Next generation EU, ma questi obiettivi, per quanto chiari, non si raggiungono indifferentemente attraverso scelte alternative molto distanti tra di loro. Non c'è un'ampia gamma di alternative intercambiabili che ci consente di avere le stesse possibilità di raggiungere quegli obiettivi. Anzi, tra le condizioni che ci consentono di raggiungere quegli obiettivi vi sono dei punti di passaggio obbligati, che portano con sé delle conseguenze sulle scelte che dobbiamo sviluppare. Mi spiego nel concreto, partendo da un dato: l'Italia, a differenza di altri Paesi, ha deciso di prendere dall'Europa tutte le risorse che era possibile prendere, sia quelle sussidiarie, e quindi i sussidi che non sono da restituire, sia quelle prestate, che rappresentano debito da restituire. Non tutti i Paesi si sono comportati come noi e questo è il motivo per il quale nella classifica delle risorse finanziarie siamo primi. Ad esempio, Germania, Francia, Spagna e Portogallo hanno scelto di prendere solo i sussidi;

La Spagna ha deciso di prendere solamente i sussidi, dicendo che intanto spenderà queste risorse e poi vedrà in quali condizioni si troverà, ed eventualmente attingerà anche alla parte a debito. Visto che abbiamo scelto di attingere a tutte le risorse e che la parte consistente delle risorse è a debito, allora c'è una parola che rappresenta un passaggio obbligato: crescita. Senza crescita non si pagano i debiti e qui il presidente Draghi ci dà un'indicazione in più, perché definisce la crescita, chiamandola crescita inclusiva. Credo che su questa definizione dobbiamo confrontarci politicamente e capirci, perché credo che la crescita inclusiva non sia da intendere in modo classico: cresciamo, produciamo *surplus* che utilizziamo per pagare i debiti, ma anche per elargire sussidi che riducono le forbici, le distanze, le differenze e le disuguaglianze.

Oggi la crescita inclusiva, per il tipo di percorso che dobbiamo fare e di cui ho detto prima, ha bisogno di un *welfare* nuovo orientato a sostenere la crescita. Anche il *welfare* deve essere un elemento di sostegno della crescita e non sarebbe neanche una novità. Facciamo un esempio. Se modificheremo - come penso - il reddito di cittadinanza - possiamo continuare a chiamarlo così - sarà per orientarlo fortemente alla formazione, di far rientrare le persone nel mondo del lavoro in modo assolutamente produttivo e adeguato alle sfide del futuro del nostro Paese. Pensiamo alla gestione delle dinamiche di transizione del nostro sistema produttivo nel nuovo orizzonte della sostenibilità *carbon free*.

non voglio ancora dire uno spartiacque, perché credo ci siano le condizioni per individuare una declinazione di questa sintesi capace di avere largo consenso e condivisione in questo Parlamento. È chiaro che la formula classica del produrre ricchezza per redistribuire oggi per il futuro è insufficiente. Almeno per me, ciò è chiaro e richiama la necessità di un profilo politico riformista.

di profilo politico riformista che ritengo sia adeguato a definire il percorso che ci porta a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati come Paese. Penso a una storica distanza dell'Italia con gli altri Paesi, che si chiama *gap* di produttività. Il presidente Draghi, anche qui, ha fissato un punto nuovo o - meglio - che necessita di un'interpretazione politica. Egli ha parlato di recupero di produttività totale dei fattori, indicatore che misura il grado di efficienza complessivo di un'economia che è diminuita del 6,2 per cento tra il 2001 e il 2019, a fronte di un generale aumento a livello europeo. Certo: noi siamo stati testimoni dell'insufficienza della definizione classica di produttività (PIL per unità di prodotto, oppure ore lavorate per unità di prodotto e anche in questo caso i grafici sono impietosi). Ma cosa è stato quota 100 se non il più grande intervento finanziato da soldi pubblici che è andato ad agire direttamente sulla definizione classica di produttività, quando i dati verificati sul campo ci dicono che, ogni dieci lavoratori che sono andati in pensione con quota 100, ne sono stati stati assunti uno o due? Avremmo dovuto registrare un miglioramento della produttività, ma questo non è successo. Ciò vuol dire che il concetto classico non descrive pienamente il problema.

giustizia, concorrenza e pubblica amministrazione sono le riforme che concorrono a far crescere la produttività del lavoro nel nostro Paese. Ne aggiungo un altro. L'articolo 46 della Costituzione recita che «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende». un articolo inattuato, un grande *gap* con l'economia forte dell'Europa, ossia quella tedesca. Voglio concludere con un'altra osservazione che credo debba essere oggetto di una riflessione urgente, come fare in modo che le risorse del PNRR rappresentino un volano per gli investimenti privati. C'è necessità di mettere questo tema in primo piano a tutti i livelli istituzionali, perché parliamo di ingenti risorse che arriveranno per gli investimenti pubblici, ma che devono rappresentare un'opportunità complessiva

in vista della legge di bilancio, contiene alcuni dettagli interessanti e positivi. È bene che il Documento rilevi che la politica è e resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la crisi, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. condizioni, secondo il Documento, saranno soddisfatte nel 2024, sebbene secondo la Corte dei conti tale previsione sarebbe potrebbe essere ottimistica, considerando - ad esempio - la nostra dipendenza dal debito pubblico. L'economia italiana, come indica il Documento, sarà certamente favorita anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quale occasione per il rilancio in chiave di sostenibilità ambientale e sociale, come sottolineato anche dalla terza del Consiglio dell'Unione europea, anche se il PNRR presenta importanti criticità proprio sulla parte ambientale, che ho a suo tempo evidenziato molte volte (e lo farò anche questa volta). È bene che venga evidenziato che le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dalla riforma dei sussidi ambientalmente dannosi andranno utilizzate

voglia di crescere e di aumentare la nostra produttività, abbiamo lasciato indietro l'ambiente. Positivi sono anche gli investimenti in ricerca, innovazione e istruzione. È in questa direzione che va orientato l'impegno di risorse pubbliche a supporto di iniziative private e, attraverso *partnership* pubblico-private, verso interventi i cui impatti sociali e ambientali siano evidenti e misurabili, con l'adozione di nuovi criteri di valutazione degli investimenti che integrino i tradizionali parametri economico-finanziari, in relazione al nuovo assetto sociale e ambientale. Inoltre, nel Documento si tratta

perché in questo caso un conto è l'ottimizzazione degli *iter* amministrativi e un conto è - ad esempio - il taglio delle consultazioni e dei termini relativi alle procedure di

nell'atto di Governo di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso delle rinnovabili. Sempre in tema di semplificazione, ricordo anche che è grave che sia stata rimandata di almeno un anno l'adozione della pianificazione delle attività marittime - è un'altra cosa della quale parlo sempre mentre si va avanti con il Pitesai, che è il Piano che riattiva le trivelle e che dà il via alla ricerca e prospezione di idrocarburi lungo le coste e le aree protette. C'erano state delle sospensioni, ma oggi si riapriranno quegli *iter* e quindi noi non difenderemo più ciò che abbiamo dichiarato nel PNRR e ciò che dichiariamo ogni volta; non stiamo facendo il *green deal*, ma stiamo facendo *green washing*. Il rischio, come manifestato anche dalla protesta dei giovani, è che tutte queste intenzioni e tutte queste misure si traducano appunto in *green washing* governativo: far vedere che si presta attenzione alle tematiche ambientali, ma in realtà poi nulla o ben poco cambia. Investire sul gas è - ad esempio - un azzardo che rischia di compromettere la transizione ecologica *(Applausi)*. E quindi noi vogliamo correre: ma dove vogliamo andare? Se infine ritengo positivo che la NADEF sottolinei la particolare importanza della mobilità sostenibile e integrata, sia di persone che di merci, e che gli investimenti pubblici dovranno contribuire contribuire a rendere il sistema infrastrutturale italiano più moderno e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione del sistema energetico, non è tollerabile che sia stato aggiunto all'ultimo momento, tra i disegni di e quindi alla prossima legge di bilancio, un ulteriore disegno di legge, di cui si è già parlato e che hanno già citato i miei colleghi con i quali ho contribuito a scrivere la proposta di risoluzione; mi riferisco al disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione. Questo disegno di legge riguarda anche l'ambiente

l'ecosistema e beni culturali. Se vogliamo cedere anche l'ambiente alle Regioni, su questo anche la riforma Cartabia ha già previsto il concerto con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e il parere della Conferenza unificata, senza considerare l'improcedibilità per i giudizi di impugnazione. Per il reato ambientale e il disastro ambientale non è prevista una proroga. Concludendo, mi asterrò dal voto perché, sebbene riscontri iniziative positive all'interno della Nota, non è stato dato al Parlamento il tempo di poter approfondire i dettagli.

essenziale per la programmazione economica e finanziaria del Paese dei prossimi anni. Al suo avvio il Governo Draghi ha dovuto affrontare una situazione caratterizzata da dati economici consuntivi e previsionali assolutamente distonici e preoccupanti rispetto a quanto analizzato nel DEF presentato lo scorso anno dal Governo Conte, dove un incauto e da noi contestato ottimismo aveva dipinto una ben più rosea realtà su cui basare la programmazione. L'attuale Governo ha saputo interpretare la situazione del contesto economico del nostro Paese in maniera più realistica e lucida, più prudenziale, e la NADEF oggi vede modificati i dati economici indicati nel DEF in modo sensibilmente positivo, mostrando una ripresa del sistema Paese che fino a qualche mese fa era insperabile. Ciò avviene grazie ai provvedimenti adottati dal nuovo Governo per consentire la ripresa del lavoro e delle attività economiche; all'ottima riuscita della campagna vaccinale - ad oggi ha coperto con almeno una dose l'83 per cento della popolazione italiana *over* 12 - al PNRR presentato nei modi e nei tempi previsti; all'autorevolezza del nostro Presidente del Consiglio in Europa e nel mondo e alla resilienza del popolo italiano. I dati economici indicano, infatti, che la crescita del PIL reale nel primo semestre dell'anno in corso ha oltrepassato le previsioni, con un rimbalzo del 6 per cento rispetto al 4,5 per cento ipotizzato dal DEF di aprile. È un dato importante e basilare per dare fiducia agli investimenti e per infondere speranza nel Paese. Fondamentali sono l'approccio e la visione che la nostra politica di bilancio adotterà nei prossimi anni attraverso una strategia di consolidamento della finanza pubblica che si baserà sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR, come gli incentivi concessi attraverso il credito d'imposta; misure che devono essere strutturali, certe e distribuite nel tempo. Servono misure che facciano da volano alla nostra economia e determinino un effetto moltiplicatore. È per questo che chiediamo la proroga del superbonus al 110 per cento fino alla fine del 2023, come quella del *bonus* facciate. il credito d'imposta per ricerca e sviluppo non sia spesso messo in discussione e fonte di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, che ne determina o meno la bontà del progetto, entrando nel merito dello stesso. Le nostre imprese e le nostre famiglie hanno bisogno di sicurezza, di regole certe, strutturali e di progettazione. Hanno bisogno anche di fare una seria programmazione per ripartire, è vero - hanno bisogno di pagare meno tasse e di avere un sistema semplificato, con meno burocrazia possibile. In questi giorni si parla di riforma del fisco. La bozza di legge delega presentata al Consiglio dei ministri ha assorbito le linee e i principi delle proposte fatte da Forza Italia per un sistema tributario più semplice, basato sulla crescita, con riduzione del cuneo fiscale, con la rimodulazione degli scaglioni dell'Irpef, la riduzione delle aliquote, il superamento dell'IRAP e, soprattutto, con la chiara intenzione del presidente Draghi di non voler aumentare la pressione fiscale. La riforma fiscale è uno dei 20 disegni di legge collegati alla legge di bilancio a completamento della manovra stessa, cui saranno collegati altri 19 disegni di legge, alcuni già avviati in Parlamento, di natura economica, finanziaria, industriale, sociale e culturale per far progredire contemporaneamente i diversi settori in un quadro complessivo di riforme. Sarà indispensabile concentrarsi sul nuovo piano per le politiche attive, che includa la revisione del reddito di cittadinanza - lo continuiamo a ripetere e non lo facciamo certo per spirito di contraddizione, perché sono i dati che ci dicono che non funziona così com'è fatto con l'adozione di un sistema che distingua il sostegno al reddito a chi ne ha veramente bisogno dalle politiche attive del lavoro, per le quali invece si deve investire in favore di formazione, aggiornamento di competenze, posizionamento e riposizionamento nel mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione risulta infatti ancora molto elevato e invariato rispetto alla previsione di aprile, che si attesta appunto al 9,6 per cento, e la previsione non è tra le più rosee nemmeno per il 2024, con un tasso ancora elevato pari al 7,7 Pertanto, si deve necessariamente provvedere anche alla riforma degli ammortizzatori sociali e a favorire l'incrocio tra domanda e offerta. Nella NADEF sono evidenziate anche criticità e incognite che non devono essere trascurate, dalla carenza delle materie prime ai forti aumenti del costo delle stesse, dall'aumento delle energie alle tensioni finanziarie in Cina e alla fragilità del settore immobiliare, che incideranno non poco sul costo delle produzioni e sul loro rallentamento. ciò che sta purtroppo avvenendo, per esempio, nel settore dell'*automotive*: secondo una società di analisi, tra il 2021 e il 2022 si rischiano di perdere 13,5 milioni di vetture in termini di produzione globale per la difficoltosa reperibilità di microprocessori, un danno dovuto alla congiuntura, che inciderebbe non poco sulla crescita dell'economia. Vi è però anche un problema a medio e lungo termine in un'ottica di transizione ecologica dettata da direttive europee che devono però tener conto della sostenibilità sociale ed economica. Per far fronte alla cessazione del motore endotermico entro 2035 si deve già partire da oggi con la produzione di auto elettriche, il che comporta una stima di perdita in Italia pari a 70.000-100.000 occupati solo nel comparto della produzione, che ad oggi vede impiegate 350.000 persone. Bisognerà quindi supportare attentamente nei tempi e nei modi la transizione ecologica; viceversa, vi saranno forti e gravi ripercussioni occupazionali ed economiche con corrispondenti conseguenze sul bilancio dello Stato. Pur non nascondendo le possibili incognite dettate anche da una dinamica della pandemia ancora in parte imprevedibile, le prospettive indicate nella NADEF delineano comunque uno scenario di crescita. Quello che ci rassicura è l'intento esplicito di dare un'impronta espansiva alla politica di bilancio, fino a quando il PIL

di quegli anni per mancanza di investimenti e sostegno al nostro sistema produttivo. È vero, l'Ufficio parlamentare di bilancio, nella sua validazione della NADEF frena l'ottimismo rispetto al calo del debito pubblico ed è per questo che bisogna correre, correre e correre con le riforme e distinguere, come ha fatto il presidente Draghi, il debito buono da quello cattivo.

come sappiamo, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è propedeutica alla legge di bilancio e registra, in buona sostanza, i più recenti effetti circa le riforme strutturali e gli interventi di politica economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni, aggiornando di conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l'anno in corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF dello scorso aprile. La Nota 2021 risulta corredata da molteplici allegati, contenenti le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Alla relazione è allegato anche un quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale. In un'apposita sezione del quadro riassuntivo è esposta la ricognizione di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. altresì corredata da un rapporto programmatico, nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate, o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ma anche quelle che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità e che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Infine, contestualmente alla Nota, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento. La NADEF 2021 prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico. L'intonazione della politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi due anni e poi diventa gradualmente più focalizzata sulla riduzione del rapporto debito-PIL. La visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024 è positiva, nonostante le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri siano legate all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale e saranno anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, nonché dalla fragilità del settore immobiliare e dalle conseguenti tensioni finanziarie che potrebbero avere ripercussioni sull'economia mondiale. Vi è dunque una concreta possibilità di recuperare gradualmente normali livelli di apertura nelle attività sociali, culturali e sportive, il che contribuirà a raggiungere il livello di PIL trimestrale pre-crisi entro la metà del prossimo anno. Conseguita questa prima tappa, comincerà la fase di vera e propria espansione economica, che porterà la crescita del PIL e dell'occupazione nettamente al di sopra dei ritmi registrati nell'ultimo decennio. Questa mia relazione, d'ora in poi, sarà focalizzata sulle indicazioni di crescita relative ai settori della cultura, della scuola, dell'università e della ricerca. In prima analisi, è in corso di approvazione definitiva un disegno di legge che semplifica le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate. Si tratta delle cosiddette lauree abilitanti, che consentono al neolaureato di poter esercitare la professione senza attendere i tempi del superamento dell'esame di Stato. Nell'ambito dell'alta formazione, alle imprese che sostengono finanziariamente, quindi tramite dotazioni, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, con un'attenzione particolare per le piccole e medie imprese. Al fine di promuovere lo sviluppo e potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute che non superino i 9.000 iscritti, è attribuito un contributo complessivo di 2 milioni nel 2021. Di conseguenza, le risorse di bilancio verranno in misura crescente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione. Per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese e di quelle che operano nel settore della filiera agricola sono stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie. Per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono stati autorizzati complessivamente 2,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2023, a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore culturale e dello spettacolo e delle imprese delle filiere agricole, della pesca, dell'acquacoltura e delle imprese armatoriali. Con riferimento ai servizi di asili nido, l'obiettivo è quello di assicurare che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire entro il 2026 del entro il 2026 del servizio su base locale. Saranno inoltre introdotte misure volte a potenziare il trasporto scolastico di studenti disabili delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per il settore della scuola, dell'università e della ricerca si rilevano in particolare le misure per contenere il rischio epidemiologico nell'anno scolastico 2021-2022 e per garantirne l'ordinato avvio e assicurare la continuità didattica. Sono state inoltre assegnate risorse per la promozione della ricerca, l'innovazione tecnologica e viene rifinanziato il fondo volto all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa e quello per gli interventi perequativi destinato a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività destinate a potenziare l'offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base e il consolidamento delle discipline. inoltre previsto un certo numero di riforme settoriali basate su modifiche normative in specifici ambiti o attività economiche per migliorarne il quadro regolatorio, tra cui in particolare una definizione dei criteri ambientali finalizzati agli eventi culturali, insieme con un pacchetto di riforme nel campo dell'istruzione che riguardano, in particolare, le modalità di reclutamento dei docenti e il sistema degli istituti tecnici e professionali, oltre che quello dell'università, con particolare attenzione alle classi di laurea e ai corsi di dottorato. Significativo sarà anche l'impegno - e per questo esprimo particolare soddisfazione per i lavoratori dello spettacolo. Mi sembra quindi opportuno sottolineare in questa sede che le Commissioni 7a e 11a del Senato hanno avviato un ampio esame per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti in favore dei lavoratori del settore. Per esempio, si istituirà presso il Ministero della cultura il Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, si amplieranno le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo e si demanderà all'INPS l'attivazione di specifici servizi proprio per i lavoratori dello spettacolo. nella NADEF è ben riportato che viene istituito il Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e 250 milioni annui a decorrere dal 2022, per promuovere lo sviluppo della ricerca di base. Mi pare quindi opportuno cogliere l'occasione di tale significativo finanziamento per complimentarmi con il fisico Giorgio Parisi, di recente insignito del premio un evento straordinario se consideriamo che dopo sessantadue anni è la prima volta che l'ambito premio viene assegnato ad un italiano che ha svolto la maggior parte del suo lavoro in Italia.

Nobel, possa contribuire a migliorare effettivamente e una volta per tutte la situazione della ricerca in Italia che ha tanto bisogno di essere sostenuta.

economia e finanza, come spesso succede a questo genere di documenti, è molto bella nella presentazione, nella narrazione narrazione e nelle previsioni (abbiamo tantissime belle previsioni), ma in quello che possiamo toccare con mano le cose sono assai diverse.

incremento del prodotto interno lordo, stimato al 6 per cento per quest'anno. Dobbiamo vedere se ci si arriverà, ma noi speriamo che sia a questo livello, perché Fratelli d'Italia è innanzitutto a favore dell'Italia, non di questo o di quel Governo; anzi, noi speriamo che sia anche di più del 6

è che addirittura il debito pubblico scende: un miracolo straordinario, annunciato molte volte nel corso degli anni e mai avvenuto, per la verità, se non molto tempo fa. Pertanto, che avvenga adesso in un periodo così difficile sarebbe veramente

Pertanto, sempre supponendo che questa previsione sia corretta, siamo ancora a meno 3,6 per cento rispetto a due anni fa. Tra l'altro, la discesa del prodotto interno lordo del 9 per cento l'anno scorso, come sappiamo bene, è sì legata alla questione della pandemia, un fatto indubbiamente al di là del controllo in sé dei Governi, ma guarda caso l'Italia è il Paese che che ha avuto il più grande calo di prodotto interno lordo di tutta l'Unione europea. E sì che ci sono ventisette Paesi, alcuni con economie deboli e in situazioni difficili che hanno anch'essi avuto un gran numero di di morti, di contagiati e di ricoverati a causa del Covid. Tuttavia, pur essendo tutti coinvolti nella stessa pandemia,

si è sicuramente riflettuto in un calo spettacolare del PIL e dunque della ricchezza del Paese, con tante aziende che sono state in difficoltà, altre che hanno chiuso o hanno spostato le loro produzioni, e ci sono stati tantissimi posti di lavoro questo di fronte a numeri della pandemia che non sono assolutamente migliori di quelli degli altri Paesi, anzi sono spesso peggiori sia per quanto riguarda la mortalità che la letalità. Un secondo aspetto di cui pure si è molto parlato è l'incredibile calo del debito pubblico del 2021. Non sappiamo come finirà il 2021, sappiamo come sono andati i primi sette mesi, e questo non da qualche organo di informazione sovversivo di opposizione o chissà cosa, ma dai dati della Banca d'Italia. Tali dati Tali dati ci dicono che nei primi sette mesi di quest'anno il debito pubblico è aumentato di 152,9 miliardi: è il più grande aumento della storia del nostro Paese; mai

che il debito pubblico scende quando è salito più di quanto sia mai cresciuto nella storia d'Italia? È possibile perché si ricorre al rapporto tra il debito pubblico e il PIL e cioè essendoci questa risalita, a seguito della disastrosa caduta dell'anno scorso, in rapporto al prodotto interno lordo previsto ci sarebbe un miglioramento in percentuale. Siccome, però, gli italiani, le aziende e anche lo Stato non pagano le cose che devono pagare in percentuale, ma in euro,

99 miliardi di ricchezza in più rispetto all'anno passato. Sono parecchi in meno rispetto a due anni fa, ma perlomeno rispetto all'anno passato sarebbe un miglioramento. Che dire, però, di questo miglioramento di 99 miliardi quando il debito aumenta di 152,9 miliardi? A me sembra un disastro.

che questo debito, se anche scende - si fa per dire - al 153,6 per cento (queste sono le previsioni) nel corso di quest'anno, due anni fa era al 134,

solo due bienni nella storia d'Italia in cui - in termini percentuali, non in termini assoluti - l'indebitamento è stato maggiore e questi due bienni sono stati il 1918-1920, cioè

del Covid) e il 1940-1942, cioè l'inizio della Seconda guerra mondiale, con tutto quello che ha significato. Questo vuol dire che in tutti gli altri bienni della storia d'Italia c'è stato un andamento migliore. Anche in

è buono, perché quando il PIL è prodotto da generose donazioni del Governo, che in qualche caso sono dovute e giuste, quando si tratta di rifondere i danni a coloro le cui attività sono state chiuse per leggi dello Stato di erogazioni di carattere assistenziale, come il reddito di cittadinanza, non è che sia tutta salute. Siamo in una situazione in cui le nostre aziende e i singoli lavoratori sono messi in gravi difficoltà da una serie di fattori,

in modo molto significativo alla decisione politica dell'Unione europea, sostenuta anche da questo Governo, di tagliare ulteriormente le emissioni di anidride carbonica,

Questo vuol dire che le nostre bollette sono destinate ad aumentare ancora. Come si fa a essere concorrenziali in questa situazione? Concludo, Presidente, dicendo che c'è un aspetto che manca del tutto: c'è un grave *deficit* che

Quando i nati nel 2020 saranno nell'età feconda, ci saranno meno nati, anche a parità di tasso di fecondità che è del tutto opinabile che resti uguale. È molto grave, e su questo nella Nota di aggiornamento al nostro esame non c'è alcunché, se non un accenno all'assegno unico universale come abbiamo già visto, in molti casi riduce sensibilmente quello che ricevono molte famiglie, mentre altre famiglie che nulla avevano continuano a non avere Signor Presidente, la Nota di aggiornamento contiene due buone notizie che vanno sottolineate,

ed è un rimbalzo che lascia l'Italia un po' più indietro, a fine 2021, rispetto al recupero della zona euro. È una ripresa molto significativa, superiore alle aspettative, ma su cui prospetticamente gravano alcune incognite, giustamente evidenziate nella Nota: la pandemia, perché i numeri dell'Italia sono positivi sia sul versante dei contagi sia sul fronte della vaccinazione - e questo va ascritto a merito del Governo e della politica di rigore che è stata seguita e che noi abbiamo sostenuto ma non siamo fuori dall'emergenza. La seconda incognita riguarda il rialzo del prezzo delle materie prime, dell'energia e di molti semilavorati, che sta rallentando la ripresa a livello globale. I numeri che il Fondo monetario internazionale nei prossimi giorni evidenzieranno una limatura al ribasso delle prospettive di crescita a livello globale, legate anche a questi fattori. Il terzo punto da guardare con attenzione in una fase di ripresa sono le ferite sociali, aperte e aggravate dalla pandemia, con cui dobbiamo fare i conti. Il 2020 ha registrato un milione di poveri in più e a luglio di quest'anno gli occupati erano ancora inferiori di mezzo milione di unità rispetto al dato pre-Covid di due anni prima, e l'80 per cento di questi posti di lavoro che mancano all'appello sono lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti che hanno cessato l'attività e che non sono stati ancora coinvolti dalla ripresa. La seconda buona notizia - oltre a una crescita migliore delle previsioni - è che i conti pubblici vanno meglio delle aspettative: il *deficit* al 9,4 anziché all'11,8 è un dato importante sul debito pubblico, che si prevedeva in aumento e a fine 2021 dovrebbe essere invece inferiore al livello del 2020. È proprio questo buon andamento dei conti pubblici che permette al Governo di impostare una manovra espansiva nel triennio, con numeri significativi superiori a un punto di PIL di differenziale programmatico tendenziale, senza chiedere al Parlamento un ulteriore scostamento, cosa che non accadeva da parecchio tempo. Questo, oltretutto - lo sottolineo - programmando nel triennio un indebitamento netto lievemente inferiore a quello che era stato programmato nel DEF di aprile: un dato che naturalmente rafforza la nostra credibilità a livello europeo in una fase di passaggio delicata, in cui si andrà a ridiscutere le regole di coordinamento economico a livello comunitario, ma che comunque va sottolineato in questa discussione. Questa manovra espansiva del Governo che dovrebbe valere in termini netti 22 miliardi nel 2022, 29 nel 2023 e 24 nel 2024, riteniamo debba caratterizzarsi fortemente per un segno di coerenza e complementarietà con gli obiettivi strategici, gli investimenti e le riforme che abbiamo scritto nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Deve farlo su due versanti. Il primo riguarda la crescita e lo sviluppo del Paese; siamo al più 6 per cento nel 2021, cresceremo in modo consistente anche nel 2022, ma la vera scommessa è è imboccare un sentiero di sviluppo molto più sostenuto rispetto alla sostanziale stagnazione che il Paese ha sofferto negli ultimi vent'anni. vent'anni. Credo che le scelte che andremo a fare nella manovra di bilancio devono essere coerenti con l'obiettivo di accelerare ulteriormente questi numeri positivi. Lo possiamo e lo dobbiamo fare sul lato della domanda, stimolando gli investimenti a partire da quelli privati. Questo chiama con sé il tema degli incentivi per l'edilizia sostenibile, a partire dal superbonus che il presidente Draghi si è impegnato a prorogare al 2023, transizione 4.0, un pacchetto di incentivi per gli investimenti delle famiglie e delle imprese di cui noi chiediamo la proroga, ma che io credo debbano essere anche riorganizzati in una prospettiva di medio periodo. La rigenerazione energetica degli edifici, così come la digitalizzazione del settore industriale, è un obiettivo di medio periodo e noi, al di là di quello che faremo per il 2023, dobbiamo dare certezze agli operatori anche di medio periodo iniziando a discutere e decidere che cosa fare dopo il superbonus e dopo transizione 4.0. Dobbiamo stimolare i consumi delle famiglie e questo rende necessaria una riflessione su cosa fare in una fase di ripresa inflazionistica. Il caro energia è un tema che non si fermerà all'ultimo trimestre del 2021 ed è necessario un intervento strutturale di spostamento sulla fiscalità generale degli oneri di sistema. È necessario affrontare il caro energia non solo per la parte più fragile della società che usufruisce del *bonus* luce e del *bonus* gas. C'è un problema di ceto medio che va tutelato di fronte alla ripresa dei prezzi dell'energia e dell'inflazione. Dobbiamo farlo anche con l'avvio della riforma fiscale, che riteniamo debba cominciare dall'Irpef e, in particolare, da un taglio del cuneo fiscale, a partire da ciò che va ad aumentare le buste paga dei lavoratori e anche da misure che agevolino i secondi percettori di reddito stimolando l'offerta nel mercato del lavoro. Dobbiamo lavorare per lo sviluppo anche sul versante dell'offerta. Il tema delle politiche industriali è affrontato nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, ma c'è tanto lavoro da fare. Dobbiamo capire chi realizzerà le opere pubbliche in un Paese in cui i grandi soggetti dell'edilizia sono ridotti ai minimi termini. Dobbiamo capire come aiutiamo turismo e commercio a riorganizzarsi dopo le perdite durissime che hanno subito nel 2020. È una ripresa ancora parziale. Dobbiamo sostenere e accompagnare verso la transizione ecologica settori rilevantissimi dell'economia italiana che saranno chiamati a profonde trasformazioni e dobbiamo decidere misure creditizie che vadano al rinnovo del Fondo centrale di garanzia. di garanzia. Dobbiamo però altresì capire come rendere sostenibile per tantissime imprese il servizio di 230 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato che hanno salvato il sistema produttivo italiano, ma che oggi dobbiamo rendere sostenibili per i prossimi anni, evitando di comprimere i margini di investimento. Il secondo versante di organizzazione della manovra riguarda il modello di sviluppo che abbiamo scritto nel PNRR su tre punti: lavoro, *welfare* e istruzione e ambiente. La riforma degli ammortizzatori sociali è centrale e dobbiamo investire sul *welfare* e sul sistema dell'istruzione, così come sul Sistema sanitario nazionale, imparando la lezione della pandemia. Il dato tendenziale sul fondo sanitario ci riporta ad un livello inferiore rispetto a quello del 2019 e lo stesso vale per la scuola. Dobbiamo invertire questa tendenza nella manovra e recuperare il *gap* che ci separa dagli altri Paesi europei. sull'ambiente, oltre alla proroga degli incentivi per gli investimenti *green* delle famiglie e delle imprese, riteniamo sia necessario un vero e proprio fondo sociale per la conversione ecologica dell'economia. Dobbiamo accompagnare e sostenere le imprese e i lavoratori, che saranno chiamati a sfide formidabili nei prossimi anni, perché la transizione ecologica è una necessità, ci crediamo, ma non sarà un pranzo di gala e la politica economica deve tenerne conto.

applicato anche alla disciplina del lavoro. Quindi, per poter accedere al luogo di lavoro, addirittura anche in *smart working*, ci vorrà il *green pass*,

sottrae alla nostra sanità pubblica ben 6,2 miliardi di euro, rispetto ai 7,4

la campagna del commissario Figliuolo, 0,7 miliardi di euro per gli incentivi ai medici vaccinatori e 0,2 miliardi di euro per la ricerca sui nuovi vaccini contro patologie infettive. che sarà un ciclo continuo e che questo Covid *business* diventerà un affare che si protrarrà per tutto il tempo necessario, affinché le *big pharma* possano ingrassare con i soldi del nostro debito. Alla sanità ordinaria, per le liste d'attesa, spettano

I medici del 118 hanno degli stipendi talmente bassi, che ormai rifiutano quel tipo di incarico e si rivolgono ad altre tipologie di incarichi, tanto che abbiamo le ambulanze demedicalizzate. La sanità in Calabria è un disastro totale, ma l'importante è che ci sia il *green pass*. È questa la sanatoria di tutti i mali, specialmente per gli amministratori locali, ovvero i Presidenti di Regione e i sindaci, che così non hanno dovuto fare nulla le misure e i protocolli di sicurezza da associare necessariamente alla pratica vaccinale e a tutte le altre pratiche. Non hanno fatto nulla e si sono

applicate attraverso il *greenpass* ai diritti costituzionali dei cittadini incideranno sulla nostra economia reale. Una famiglia normale dovrà scegliere se pagarsi i tamponi oppure andare al ristorante. *(Applausi)*. Penso che sceglierà di pagarsi i tamponi e non di andare al ristorante. Peraltro, pagarsi i tamponi per evitare

né l'informazione *mainstream* che siamo costretti ad ascoltare tutti i giorni, con toni che rischiano di far scoppiare a breve una guerra civile. Ciò che state facendo è veramente grave,

le soluzioni del Governo dei migliori? A questo punto, non ho null'altro da aggiungere.

con l'approvazione della NADEF ci sia qualcuno, come il sottoscritto, che dica che c'è anche un po' da preoccuparsi.

crescita, che è molto forte, in controtendenza rispetto alle altre economie europee, però dico che un po' ci dobbiamo preoccupare. Non mi dispiaccio del fatto che il rimbalzo del nostro PIL sia positivo, ci mancherebbe, ma dobbiamo pensare che

che questa crescita è dovuta alla capacità delle nostre imprese di riprendere il lavoro e di conquistare i mercati, specialmente quelli internazionali, aiutata sicuramente dalle dalle manovre espansive adottate a livello nazionale e comunitario. Dobbiamo pensare che questa nostra crescita è dovuta anzitutto alle nostre eccellenze produttive. Quest'anno poi siamo eccellenti in tutto: nello sport abbiamo vinto di tutto,

alla politica della BCE, che sta tenendo i tassi di interesse su livelli molto bassi (come non lo sono mai stati), e alle scelte di Bruxelles, che ha sospeso qualsiasi politica di rigore nei bilanci dei singoli Stati attraverso il *temporary framework* e ha varato il *recovery plan*, che farà arrivare all'Italia oltre 200 miliardi, che porteremo a terra attraverso il PNRR. Queste sono due precondizioni fondamentali, però - ed ecco i motivi di dubbio

con la politica di sviluppo, anche ecologico, che nel prossimo futuro sarà un potente fattore di crescita. Con l'approvazione della il Governo ci offre una cornice macroeconomica rispetto alla quale sono già indicate le future politiche di bilancio, cioè come si evolverà la tassazione se saranno spesi bene i soldi. Partiamo da alcuni capisaldi chiari: la situazione è migliore di quella prevista la scorsa primavera,

L'ambizione è di mantenere una crescita elevata anche per i prossimi due o tre anni, perché solo in questo modo potremo puntare a dare lavoro a quanti lo hanno perso e ai tanti giovani che non l'hanno avuto (si tratta di oltre 3 milioni di cittadini). Se vogliamo arrivare vicini alle percentuali di impiego degli altri Paesi europei, europei, non bastano gli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati dall'Europa, ma ci vogliono cambiamenti nel nostro modo di essere, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dalla scuola al mercato del lavoro, alla formazione professionale verso le nuove tecnologie.

quota 100, per certi aspetti, e il reddito di cittadinanza. È mai possibile che siano allocati 10 miliardi per il reddito di cittadinanza e 3 per sostenere le imprese in crisi in questo momento? *(Applausi)*. C'è un tema che emerge e che abbiamo posto anche stamattina nell'audizione con il signor Ministro. Non è che ci preoccupa solo l'aumento del costo energetico; ci preoccupa il costo esponenziale impazzito delle materie prime: non se ne trovano più e le nostre imprese - come dicevo stamattina rischiano di chiudere e di fermare le commesse, perché non arrivano materie prime. Secondo argomento: non si trova manodopera. Interi settori del nostro Paese, nel terziario e nel turismo, non riescono a offrire servizi di un certo livello, perché non si trova personale.

disegni di legge collegati alla NADEF, che saranno allegati, perché da lì si capirà seriamente se il Governo avrà intrapreso definitivamente la strada giusta. C'è un cronoprogramma da mal di testa, secondo me, tanti e tali sono gli argomenti: diamo quindi il nostro appoggio al Governo e al presidente Draghi, vera eccellenza del nostro Paese in questo momento, e non stanchiamolo con le nostre sterili polemiche, perché il Paese ha bisogno di un uomo come lui!

È una legge chiara: c'è un disegno macroeconomico che, se va avanti così, porta la gente che sta male a stare peggio e quella che sta bene a stare meglio. Se questo è il disegno di società che vogliamo, perché non possiamo toccare i mostri sacri come reddito cittadinanza e quota 100, diciamo fin da subito che non ci stiamo,

ho fatto un esercizio che penso possa servire anche alle poche persone che stanno

Sono tornata indietro e mi sono guardata la NADEF del 2019, perché avevo necessità di riuscire a comprendere anche il documento che ci è stato consegnato

a parte i concetti più volte giustamente ribaditi - la congiuntura dell'economia italiana si fermi a un livello di previsione nel 2022,

Leggo brevemente le prime dieci righe della NADEF del 2019, che sono le parole della relazione dell'allora ministro Gualtieri: «Negli ultimi quindici mesi l'Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti turbolenze internazionali si sono assommate ad un'accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti. Il nuovo Governo si è da poco insediato in un contesto di bassa crescita e persistente disagio sociale. Nonostante le misure importanti adottate negli ultimi tempi, le disuguaglianze all'interno della nostra società restano acute e le sfide che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciononostante, la resilienza che l'Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario ed istituzionale fornisce una solida base di partenza In questo contesto, l'Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo (...). La bassa crescita dell'economia italiana è il portato di problemi strutturali ormai di lunga data».

che sta dispiegando la propria efficacia. Ciò ha consentito di attuare le restrizioni imposte alle attività produttive. I dati sulla pandemia restano tuttavia molto elevati.

bilancio va avanti dunque con la stessa identica metodologia ed è giusto, perché è quella che viene adottata per la validazione di questo documento, che viene poi portato all'attenzione del Parlamento.

ne sono alcune che hanno necessità di correre molto più velocemente di altre, altrimenti, quando sarà ora di usare questi soldi, ci troveremo completamente fermi.

Questo comporta ovviamente che quelli che sono al di fuori di quest'Aula abbiano un filino di paura, paura, dagli imprenditori al semplice cittadino: l'imprenditore, l'artigiano, quello che ha il negozio che vende il pane, quello che ha il supermercato o il benzinaio si chiedono come sarà la situazione, cosa succederà e quali saranno le riforme. un po' di certezza, non solo nei tempi, ma anche nei contenuti, perché, se non diamo certezza nei contenuti a quelli che stanno fuori, oltre a non capire il perché si rimutuano in continuazione dopo anni, anche se si capisce tranquillamente leggendo...

da farci arrivare, magari nel 2022, a dire di non aver avuto una grande crescita, ma che non c'è una decrescita, che finalmente la diseguaglianza si è un pochino attenuata, il sistema dei trasporti è migliorato,

vorrei concentrarmi sui numeri contenuti all'interno di questa Nota di aggiornamento del DEF per quanto riguarda la sanità, il nostro scudo nei confronti dell'emergenza e della pandemia. In questa NADEF si parla di rafforzamento del Servizio sanitario nazionale

I numeri di questa NADEF, del Fondo sanitario nazionale, sono di un 7,5 per cento rispetto al PIL nel 2020, che scende al 7,3 nel 2021, per poi scendere ulteriormente al 6,1 negli anni successivi. Nominalmente però la questione per fortuna è un po' diversa, perché partiamo da 123 miliardi nel 2020, saliamo a 129 miliardi

il rapporto rispetto al PIL era sempre stato intorno al 6,6 per cento, quindi ci auguriamo che anche nei prossimi anni ci sarà un aggiustamento in quella direzione, per non scendere al di sotto di tali livelli. Una flessione è comunque attesa e la auspichiamo tutti, perché per esempio circa 7 miliardi dei 129 spesi in questo 2021 sono a fronteggiare la pandemia, riguardano i vaccini, le spese della struttura commissariale per l'emergenza, i fondi per la somministrazione dei vaccini e l'abbattimento delle liste d'attesa che si sono allungate nel periodo in cui i nostri ospedali hanno dovuto far fronte all'emergenza Covid e non hanno potuto espletare tutte le prestazioni routinarie che avevano sempre fatto. Di fianco ai fondi stanziati all'interno del nostro bilancio, ci sono poi quelli che arriveranno dal PNRR, come i 15 miliardi della missione 6: missione 6: verranno spesi per cambiare la nostra medicina territoriale e far fronte alle criticità emerse durante la pandemia, ma che io e i miei colleghi in 12a Commissione avevamo evidenziato già precedentemente e che solo un'emergenza mai vista prima nel nostro Paese e nel mondo è riuscita a far balzare agli onori della cronaca e a rendere evidente a tutti, anche all'interno di quest'Aula.

e stretture delle norme che impediscono di far fronte alle carenze, come hanno fatto fino ad ora. Ci siamo resi conto che avevamo bisogno di più medici, di più infermieri, di più operatori sanitari

una valorizzazione dell'esperienza di questi precari, perché hanno acquisito competenze, conoscenze e professionalità sul campo e non possiamo dimenticarcene da domani, quando speriamo che l'emergenza Covid sia finita. dicendo che il PNRR prevede la riforma della medicina territoriale, perché tutti abbiamo visto che è mancata in tantissime Regioni la figura del primo contatto per i cittadini sul territorio. Ci sono state difficoltà nel rapporto con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta,

di lavoro e il loro rapporto di collaborazione col Servizio sanitario nazionale. *(Applausi)*. Vanno inquadrati diversamente: valutiamo come quale sia il modo migliore, ma bisogna sicuramente cambiare qualcosa, perché qualcosa certamente non ha funzionato. Da circa un anno la 12a Commissione sta affrontando un affare assegnato proprio sulla medicina territoriale e su quello che dovrà essere nell'epoca *post*-Covid.

da un punto all'altro del nostro territorio, come diversi sono stati le prestazioni e il modo di affrontare la pandemia. Bisogna che anche queste figure abbiano una specializzazione universitaria, che garantisce più uniformità, più qualità e più qualificazione per chi esce da tale formazione. Bisogna che rafforziamo la figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, che abbiamo introdotto già l'anno scorso, ma non a sufficienza. Abbiamo visto infatti che, nei territori in cui questa figura già esiste, è molto utile all'insieme della medicina territoriale: riesce a seguire meglio i pazienti a domicilio (cosa che dovremmo fare sempre più nei prossimi anni); a limitare gli accessi dei cosiddetti codici bianchi ai pronto soccorso; riesce quindi a dare una risposta al bisogno di salute dei cittadini. Tale risposta non può essere a macchia di leopardo sul territorio nazionale: quello che ci ha insegnato questa pandemia, che già qualcuno sapeva e cercava di gridare inascoltato, è che la sanità dev'essere uguale dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, perché è inaccettabile che non ci siano le stesse prestazioni e gli stessi bisogni esauditi dovunque sul nostro territorio. Con i fondi del PNRR e con le risorse che stanzieremo nei prossimi anni dobbiamo fare in modo che tutte queste disuguaglianze vengano annullate e che gli stessi diritti siano esigibili ovunque.

nel passato, perché bisognava potenziare la medicina territoriale. Quest'ultima non era stata potenziata dappertutto e, adesso che lo faremo, non cerchiamo però di fare risparmi sempre utilizzando la sanità quasi fosse un bancomat come in passato, riducendo ancora le prestazioni ospedaliere, perché sono già al livello minimo. Cerchiamo quindi di non sbilanciare dall'altra parte il nostro sistema sanitario. Non dimentichiamo una cosa importante, accaduta durante questa pandemia: mi riferisco al bisogno di far fronte anche alle esigenze della salute mentale. Non posso dimenticare quello che mi ha detto una collega ieri, riguardo all'alto tasso di suicidi nella sua città e nella sua Regione, soprattutto tra gli adolescenti. Abbiamo svolto un affare assegnato con la 7a Commissione proprio sul modo in cui i giovani e gli adolescenti hanno affrontato la pandemia, come si sono rapportati con la didattica a distanza, e abbiamo visto che i più fragili hanno riportato le conseguenze peggiori. Avevamo già stanziato fondi per un supporto psicologico ai nostri ragazzi, ma nel concreto non si è arrivati ad avere dappertutto figure di supporto ai nostri studenti, quindi vigiliamo e facciamo in modo che le Regioni mettano in pratica le linee di indirizzo impartite dal Parlamento. non solo per oggi, ma anche per il futuro, perché la fragilità dei nostri giovani l'abbiamo conosciuta oggi, ma ha radici più profonde di quelle venute fuori con il Covid. Un'altra parte importante del *puzzle* nella medicina di domani sarà l'emergenza-urgenza territoriale. L'anello di raccordo tra la medicina territoriale e i nostri ospedali va rivisto: tutti gli operatori del settore dicono che non funziona ci sono criticità. Ci stiamo lavorando, ma dobbiamo fare il massimo perché anche questo pezzo del *puzzle* vada al suo posto e svolga la sua funzione nel migliore dei modi, valorizzando tutte le professionalità che ci lavorano.

perché quello che conta sarà essere in ogni modo preparati ad affrontare la futura emergenza, qualunque essa sia.

Da una parte, il tessuto produttivo ha dato grande prova di resistenza e di resilienza e ha messo in campo una straordinaria voglia di ripartire; dall'altra, bisogna dire che questo Governo ha creato le condizioni affinché ciò accadesse, alla campagna vaccinale e alla saggezza con cui sono state gestite le riaperture, ma anche all'idea di un Governo che infonde fiducia nei cittadini, perché si concentra sulle questioni reali. Sappiamo però che non mancano le incognite. Innanzitutto, spero davvero che l'estensione del *green pass* ai luoghi di lavoro sia sufficiente per dare il colpo di coda alla campagna vaccinale, raggiungendo quanto prima l'immunità di gregge,

Vi è poi il problema internazionale delle materie prime, a cominciare dalle forniture energetiche. Gli interventi previsti dal Governo affrontano la questione, ma è evidente che ci sarà comunque un contraccolpo sulle famiglie e sulle imprese. anche il problema legato alla crescita dell'inflazione, collegato sia alla questione delle materie prime, sia al rimbalzo economico internazionale. È importante quindi che queste problematiche vengano affrontate per proteggere la crescita del PIL. Un'altra questione a cavallo tra presente e programmazione è il tema occupazionale. Siamo in uno strano paradosso: da una parte, segniamo livelli di crescita per la prima volta sopra la media europea; dall'altro, si perdono posti di lavoro; da un altro ancora, c'è una difficoltà a reperire lavoratori qualificati nei servizi, nell'artigianato e in altri settori.

la pandemia ha messo a nudo tutti i ritardi e i limiti del nostro mercato del lavoro. Il tasso di occupazione basso è quindi una delle radici del problema della poca crescita negli ultimi vent'anni, dai limiti del nostro mercato del lavoro. Occorre, quindi, una riforma che nel contesto di un rafforzamento degli ammortizzatori sociali renda più dinamico l'incontro tra domanda e offerta. Al contempo, occorre un massiccio intervento sulle politiche attive, su una formazione davvero connessa con il mondo del lavoro, e su politiche di conciliazione famiglia e lavoro efficaci. occorre altresì una nuova politica per il rimpatrio dei giovani che vivono all'estero, partendo dagli ambiti accademici ma abbracciando tutte quelle professionalità di cui oggi avvertiamo carenza. Sulla programmazione questa Nota di aggiornamento pone l'accento sulle politiche fino al 2024, e tuttavia bisogna lavorare fin da adesso anche sul dopo, come creare, cioè, le condizioni per tenere assieme crescita e politiche di bilancio. Il nostro debito pubblico, cresciuto a dismisura durante la pandemia, rischia di non essere interamente sostenibile quando verranno meno tassi di interesse così bassi e l'ombrello della BCE. È vero, come ha ricordato il Ministro, che il 2022 è l'anno del picco del rapporto debito-PIL e che poi comincerà la fase di decantazione, ma il tema è come creare condizioni interne liberate il più possibile dalle variabili internazionali, affinché dopo il 2024 l'Italia non torni a una crescita inferiore alla media UE UE e torni, invece, a una stagione di bilanci e avanzi primari. Meno debito, in effetti, vuol dire più autonomia per l'Italia a definire le proprie politiche di bilancio e politiche economiche in generale. Qui c'entrano naturalmente le politiche strutturali: dalla riforma della giustizia, dopo la legge delega, a quella del fisco alle semplificazioni a quella del mercato del lavoro,

C'entra molto anche la capacità di investire sulla ricerca e sullo sviluppo, come ha ricordato ieri il premio Nobel alla fisica Giorgio Parisi. In conclusione, Presidente, penso che siamo sulla strada giusta, che abbiamo un quadro decisamente migliore di quello che si prospettava un anno fa; possiamo, poi, discutere di elementi di contesto - ad esempio, credo che la reintroduzione del *cashback* non sia una priorità e che sul 110 per cento bisogna sfoltire le norme e dilatare i tempi di rendicontazione e di consegna d'opera per contrattare la lievitazione dei costi di intervento ma quello che più conta è lavorare sulla prospettiva, sulla rimozione degli elementi che hanno fatto dell'Italia il Paese con la crescita più bassa degli ultimi venticinque anni tra i grandi Paesi occidentali. È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

che registra decisi miglioramenti della nostra economia, sicuramente dettati dalla ripresa delle attività, resa possibile - lo ribadisco - dalla rimozione delle restrizioni sociali e dalla grande consapevolezza, dimostrata dalla maggioranza degli italiani, rispetto alla vaccinazione e all'utilizzo del *green pass*. Questi sono veramente i presupposti sulla base dei quali l'economia può riprendere ed essere rispondente alle previsioni che la NADEF riporta a tutti noi. Il sostegno economico non è mancato a partire dal 2020 ed è stato via via crescente e più mirato alla crescita, e la NADEF lo conferma: c'è stato un rimbalzo deciso di 1,2 punti percentuali del PIL,

essa si basa su un sistema complesso e proprio l'uscita da questa crisi lo dimostra. lo dimostra. Sul lato dell'offerta lo dimostra la resilienza mostrata dall'economia nei settori dei servizi, dell'industria e delle costruzioni, sicuramente sospinta dalla misura del 110 per cento che, come annunciato, verrà prorogata, anche se non resa strutturale. Lo dimostra altresì anche il supporto dal lato dei consumi; le famiglie e le imprese hanno reagito molto bene, mettendo a disposizione il loro tasso di risparmio accumulato durante la pandemia, e le imprese, nel settore pubblico e nel settore privato, supportando la crescita economica con una grande propensione agli investimenti. Non dobbiamo dimenticare che molta parte degli investimenti è finanziata con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La metà degli investimenti previsti al 2024 sarà finanziata dal Piano di ripresa e resilienza. Questo ci obbliga a una riflessione sull'importanza strategica dell'effettiva, completa, totale ed efficace realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza perché la NADEF poggia scommette sulla crescita del PIL come chiave per risolvere la crisi e riportare anche l'indebitamento verso l'obiettivo di medio termine. Certo, ci sono altri fattori di rischio; uno fra tutti, vale la pena sottolinearlo, è stato il tema del rincaro delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti, ma anche e soprattutto del settore energetico, con particolare riferimento al gas. Nelle previsioni della NADEF l'inflazione ha un rialzo nei primi tre mesi all'1,2 e, su base annua, all'1,5

fa la dichiarazione del presidente Draghi rispetto a un centro di stoccaggio europeo del gas; mi sembra che tali soluzioni vadano nella direzione giusta per tutelare l'Europa nel suo complesso. Il quadro macroeconomico tendenziale quindi, a misure invariate, migliora sul lato PIL e dell'indebitamento netto dell'indebitamento netto che si ripropone su un percorso di riduzione fino ad arrivare sul lato tendenziale al 2,1 per cento nel 2024. Di conseguenza anche il rapporto debito-PIL si riporta più velocemente di quanto previsto nella NADEF su un percorso di riduzione che lo vede ai livelli pre-crisi, a partire dal 2030. partire dal 2030. Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico è interessante perché ci dà il respiro verso il futuro. Da questo punto di vista è molto chiaro che i prossimi due anni continueranno a essere supportati da una politica espansiva di dare il giusto supporto a famiglie, imprese e al volano del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma che essendo noi soggetti ad obblighi che torneranno in vigore a livello europeo, ovviamente in modo diverso rispetto a quelli che conosciamo sul Patto di stabilità e crescita, dovranno riportarci politiche più neutre a partire dal 2024 e, dagli anni successivi, a una maggiore attenzione sulla riduzione del rapporto debito PIL e sulla generazione di avanzi primari. Sul fronte degli avanzi primari mi preme dire che è vero che bisogna tenere sotto controllo la spesa corrente, che dovrà esserlo in rapporto ai nuovi investimenti che genereremo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovranno essere a loro volta sostenuti. vorrei poi rilevare un aumento delle entrate grazie alla lotta all'evasione fiscale. Su questo punto mi piacerebbe sottolineare che la vera lotta all'evasione fiscale è il sommerso; la finalità non dovrebbe essere il gettito, perché avere come finalità il gettito vuol dire colpire l'emerso. È troppo facile controllare l'emerso. Sicuramente va fatto, la *compliance* deve essere migliorata, ma la vera sfida dell'Italia sul lato dell'evasione è un *intelligence* sul sommerso, risparmi di imposta anche a disposizione di una pressione fiscale più bassa. Sul lato del *deficit* mi preme dire che il *deficit* programmatico è maggiore di quello tendenziale di oltre un punto percentuale su tutto il prossimo triennio e che questo maggior *deficit* verrà messo a disposizione di nuove politiche che disegneremo nella prossima legge di bilancio e che già nella risoluzione che ci apprestiamo ad approvare sono tratteggiate.

che la spinta favorevole delle politiche monetarie e finanziarie, la riattivazione dell'ottimismo dei consumi e anche la grandissima opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza costituiscano sicuramente un fattore positivo.

dell'Assemblea e del Governo deve esserci un attento monitoraggio dei rischi, perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza costituisce la vera, unica e ultima grande occasione dell'Italia e non possiamo assolutamente permetterci di sbagliare l'applicazione, l'implementazione e la realizzazione delle opere, delle riforme e del progetto politico di riassorbimento delle disuguaglianze previsto nel PNRR. Signor Presidente, che servano delle precondizioni sociali. Il clima di stabilità nazionale ed europeo in questo senso aiuta, credo però ci sia la necessità di un buon Governo, saggio e lungimirante, anche la necessità di un fortissimo radicamento europeo. Siamo nel solco di un progetto che non riguarda solo noi, ma che è molto più ampio e che la Conferenza sul futuro dell'Europa sta delineando. Questa è la direzione verso la quale l'Italia deve guardare, per tornare ad essere veramente forte e noi tutti godere del benessere di cui abbiamo avuto conoscenza in altre fasi della nostra vita. Signor Presidente, il nostro voto sarà pertanto favorevole.

di opposizione, sempre in modo propositivo, di chiarire bene questo aspetto legato agli estimi catastali. Quindi, immaginiamo e auspichiamo ci possa essere, in qualche modo, un riscontro positivo dopo che sarà ufficiale la presenza di questo nostro

in riferimento ai modi e ai tempi per approfondire questi temi, che sono sempre molto risicati, così come ha detto il mio collega, senatore De Bertoldi. Ho sentito anche i colleghi della Lega che hanno

per l'approvazione del documento. Constatiamo quindi, con molto rammarico, il ruolo sempre più marginale del Parlamento, che viene ridotto ad un'appendice del Governo, quando invece dovremmo essere in una Repubblica parlamentare, in cui il Parlamento è sovrano, in quanto espressione del popolo.

per cento su base nominale e una previsione più rosea addirittura rispetto al 5,6 per cento. Leggiamo anche del prodotto interno lordo in netta crescita fino al 2024, quando si attesterà all'1,9

numeri si scontrino con una diversa realtà che riscontriamo sul territorio. La verità è che negli ultimi due anni il debito netto è aumentato di circa 20 punti percentuali e oggi ci stiamo solo sforzando di non mandare l'Italia al collasso. Quel che più ci dispiace constatare è che i numeri di cui oggi vi vantate sono solo il sintomo di una ripresa che arriva in ritardo e non per meriti vostri, ma per la forza del popolo italiano, che non è abituato ad arrendersi nonostante voi l'abbiate abbandonato a se stesso. Queste vostre previsioni ottimistiche nascondono il fatto che se siamo in questa situazione è per colpa dei Governi che negli ultimi due anni hanno gestito l'emergenza e sprecato miliardi in mancette e prebende, in spregio alle vere e reali esigenze del Paese. Paese. Questo spreco di denaro non è una tesi inventata da Fratelli d'Italia. Persino il Capo dello Stato ha richiamato le Camere a un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione di urgenza e al rispetto dei limiti di contenuto dei provvedimenti emanati. Tradotto in parole povere, viene messo nero su bianco quello che Fratelli d'Italia denuncia da sempre. In tutti i provvedimenti emergenziali adottati negli ultimi anni sono stati inseriti commi e misure che con l'emergenza Covid nulla avevano a che fare finanziati con risorse in *deficit*. Si tratta dello stesso debito che oggi voi vi vantate di ridurre (e meno male, ci verrebbe da dire). Va anche ricordato che le vostre previsioni ottimistiche sono legate all'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che si basa su riforme di cui conosciamo ancora poco e quel poco di cui siamo a conoscenza non ci fa sicuramente dormire sonni tranquilli. Pensiamo alla riforma del fisco, sulla quale ci pare di capire che state già litigando, tanto per cambiare. Abbiamo denunciato come dietro questa riforma si nasconda una profonda revisione

anche se ieri il presidente Draghi ci ha rassicurato dicendo che il contribuente non si accorgerà di nulla. Ce lo auguriamo convintamente. Abbiamo sentore che dietro le vostre belle parole e previsioni ottimistiche si nasconda il vuoto totale. Parlate di ridurre l'Irpef e le tasse sul lavoro, ma ieri la Corte dei conti ci ha detto in audizione che non ci sono le risorse per farlo. Basate tutto sull'utilizzo delle risorse del PNRR, ma di fatto ancora non ci sono gli strumenti che consentono al Piano nazionale di ripresa e resilienza di essere efficace ed efficiente. Dite che la ripresa è dovuta anche all'incremento della campagna vaccinale, ma dimenticate di mettere in sicurezza quei luoghi dove il contagio è più facile, con o senza vaccino, tipo i mezzi di trasporto pubblico o le scuole. Vi vantate di un'occupazione che aumenta, senza tener conto del fatto che si tratta di contratti a termine e di dati inferiori al periodo pre-pandemico. A proposito di lavoro, continuate a difendere questo benedetto reddito di cittadinanza, che di posti di lavoro ne ha creati ben pochi rispetto alle vostre stesse aspettative. In pratica, fate solo tanta confusione quando gli italiani vi chiedono fatti e concretezza. Proviamo ancora una volta a chiedere interventi concreti e veritieri per le famiglie e le imprese italiane. Con la risoluzione di oggi chiediamo al Governo di impegnarsi a varare una riforma fiscale che riduca veramente gli oneri che gravano su imprese e famiglie. Pensiamo, in particolare, al cuneo fiscale, che le tasse sul lavoro rappresentano il maggior ostacolo alle assunzioni da parte delle aziende italiane. Non c'è niente di impossibile, basta eliminare il reddito di cittadinanza che vale miliardi di euro l'anno e utilizzare le risorse liberate per finanziare una vera e significativa riduzione del costo del lavoro. Chiediamo anche di non includere nella delega fiscale - come ho già anticipato - la revisione degli estimi catastali e nessuna altra misura che si possa tradurre in un prelievo legato ai beni immobili, in un momento storico così grave di crisi economica per lo Stato nazionale. Vorremmo che questo Governo iniziasse finalmente a finanziare le politiche attive sul lavoro, superando il decreto dignità e assumendo delle misure che vadano nella direzione del principio "più assumi e meno paghi". Chiediamo anche nuove misure a tutela dei lavoratori autonomi, a completamento di quelle recentemente emanate e fortemente volute dal nostro Gruppo parlamentare. Infine, dal Governo pretendiamo interventi concreti - come diceva il collega Malan prima di me - per ridurre il costo dell'energia, affinché non gravi sulle famiglie, viste le recenti notizie che annunciano forti rincari sulle bollette. Su questi punti e sugli altri contenuti nella nostra proposta di risoluzione, che per ragioni di tempo evidentemente non cito, Governo e maggioranza possono contare sul pieno appoggio del nostro Gruppo parlamentare. Per questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia sulla proposta di risoluzione accettata dal Governo sarà un voto contrario. Signor Presidente, affrontiamo oggi uno dei passaggi più importanti del ciclo di bilancio. Come sappiamo bene, la NADEF descrive la situazione economica e di finanza pubblica e fissa i paletti dell'azione programmatica dell'Esecutivo, a partire dalla legge di bilancio. I colleghi Misiani, Collina e Fedeli hanno già indicato diverse proposte del Partito Democratico verso la predisposizione della legge di bilancio, ma anche misure importanti per contrastare le incertezze possibili che possono rallentare o frenare il quadro di crescita economica che la NADEF ha validato. Dunque non le riprendo, ma senza dubbio la proroga dei *bonus* energetici per favorire il sostegno alla ripresa e alla ripartenza del comparto delle costruzioni e dell'edilizia è un elemento fondamentale per sostenere la transizione ecologica sostenibile e per metterci nelle condizioni di realizzare una conversione in chiave ecologica della nostra economia. La riduzione delle emissioni in atmosfera è una componente essenziale per far tornare i conti anche di un saldo ambientale positivo, necessario per sostenere la nuova crescita. Ma insieme a questi sono stati evidenziati tanti interventi: misure importanti per contrastare il caro energia, una delle componenti che nella dimensione globale può rallentare la crescita, insieme a diverse proposte di riforma, in modo particolare degli ammortizzatori sociali, così importanti per allineare domanda e offerta. Tuttavia il contesto è positivo. La crescita acquisita nel secondo trimestre è del 4,7 per cento, la crescita prevista e validata dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel 2021 è del 6 Il fabbisogno di cassa della pubblica amministrazione, l'andamento economico, le entrate fiscali, l'andamento dell'occupazione, il costo del debito presentano tutti tendenze migliori rispetto alle aspettative. C'è fiducia nell'Italia; la fiducia cresce e ritorna in modo particolare, in maniera così energica, grazie innanzitutto alle vaccinazioni. Il piano di vaccinazioni si rileva la più importante misura economica per sostenere la crescita. La NADEF, come abbiamo visto, non solo non prevede nuovi scostamenti, per salvaguardare la natura espansiva del bilancio (che si conferma una legge espansiva, favorevole a sostenere la crescita), ma non incorpora nemmeno eventuali nuove possibili restrizioni per effetto di possibili nuove varianti pandemiche. Dunque - lo dico con grande chiarezza e franchezza - la fase politica che abbiamo di fronte non è compatibile con le ambiguità. La fiducia delle famiglie e delle imprese è una componente essenziale per sostenere la ripresa economica. Lo dico con grande franchezza, perché le nostre libertà, in modo particolare quelle alle quali si fa riferimento ogni tanto (dimenticandoci che esiste nel concetto di libertà anche una responsabilità comunitaria nella tenuta e nell'interesse generale del nostro Paese), si realizzeranno solo con l'incremento delle vaccinazioni. È una sfida che riguarda l'Italia, ma anche l'Europa nei confronti dei Paesi meno sviluppati. Il quadro macroeconomico in questo contesto ha una delle incertezze più ampie, cioè il rischio che un terzo della popolazione globale non vaccinata possa introdurre elementi e varianti incompatibili con la tenuta del sistema di protezione che i vaccini rappresentano. Dunque, evocare le libertà individuali senza perseguire una responsabilità comunitaria è un virus da estirpare. Noi lo dobbiamo anche per rilanciare la nostra democrazia, altro che perdere tempo ad accarezzare il consenso con presunti e finti sostegni ad azioni no vax. Questo quadro economico richiede responsabilità, serietà, velocità dell'azione di Governo, capacità di mettere in protezione il Paese, anche di fronte a eventuali ritorni pandemici. Solo così riusciremo a rafforzare il quadro economico macroeconomico così importante per togliere rabbia e speranza e produrre la certezza di una crescita che sarà certamente inclusiva se sarà nelle condizioni di rimuovere le incrostazioni e gli ostacoli che ci rallentano. ci rallentano. Serve la responsabilità e non i no vax o no *tax*, come qualcuno vuole far emergere. Serve la riforma fiscale per abbassare la pressione fiscale al lavoro, alle famiglie e alle imprese; servono le riforme. Non è la stagione dei no o dei «me ne frego» nei confronti della responsabilità nazionale alla quale siamo chiamati a rispondere. *(Applausi)*. Questa è la misura e l'identità con la quale il Partito Democratico intende affrontare questa discussione. Sappiamo tutti - lo ha ricordato il Presidente del Consiglio e noi siamo d'accordo - che la sostenibilità del debito pubblico dipende dalla crescita: sarà la crescita economica che determinerà la sostenibilità del nostro debito e la capacità del nostro Paese, come abbiamo visto, ad accrescere le esportazioni, ovvero la capacità di produrre quegli elementi fondamentali e decisivi per creare lavoro.

durante la fase pandemica sono diminuiti i consumi e sono aumentati i risparmi delle famiglie e delle imprese. Oggi, solo attraverso la fiducia delle famiglie e delle imprese potremo rilanciare gli investimenti, e anche i consumi interni richiedono una misura adeguata a perseverare il concetto di fiducia nel nostro Paese. Il concetto di fiducia si accompagna al concetto di responsabilità nell'azione di una maggioranza e di sostegno al Governo per realizzare le riforme fondamentali finalizzate a cambiare le incrostazioni che rallentano la crescita. Abbiamo sempre detto che per il Governo era importantissimo attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La NADEF incorpora nei saldi di finanza pubblica l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

riformando il pilastro del *welfare*, rinunciando a ipotetici modelli di sviluppo oggi condannati alla preistoria. Non ci sarà più una crescita possibile lasciando correre sempre più forte chi già corre forte, per poi produrre le risorse necessarie per aiutare chi non ce la fa. La crescita sarà inevitabilmente nuova proprio perché sarà inclusiva. Perché sia così occorre realizzare le riforme strutturali che abbiamo di fronte. Non ci sarà crescita inclusiva se non mettiamo mano subito alla riforma degli ammortizzatori sociali, perché c'è un divario enorme tra domanda e offerta. Dovremo spostare risorse

secondo elemento fondamentale è che dobbiamo rimuovere i divari, gli ostacoli e le incrostazioni che tengono l'Italia tra i Paesi nei quali il tasso di disoccupazione giovanile e femminile è sicuramente fuori dai livelli degli Stati che guidano l'Europa. Ridurre i divari e affrontare politiche di genere è essenziale in questo contesto, è decisivo per questa nuova crescita. L'Italia deve tornare ad avere parametri di occupazione giovanile e femminile tra i Paesi più avanzati, perché solo così garantiremo strutture a questa crescita. Insieme a questo, lo dico con grande chiarezza, l'appuntamento più importante, anche per consolidare il nuovo volto dell'Europa, sarà determinato inevitabilmente dalla riforma del Patto di stabilità: lo dico al Governo, lo dobbiamo detto questa mattina al Ministro, dobbiamo prepararci a questo appuntamento. È indispensabile conoscere le priorità dell'Italia per riformare il Patto di stabilità europeo, per condannare alla storia la fase europea dei tagli lineari e per costruire una fase che sostenga gli investimenti, che ci metta nelle condizioni, a prescindere dalle norme europee, di rilanciare gli investimenti, perché la crescita sarà strutturale solo nel rilancio degli investimenti pubblici e privati. Decisiva sarà la riforma del Patto di stabilità. Noi abbiamo fiducia - lo dico con grande chiarezza - nell'azione del Governo Draghi. È per questo che oggi voteremo favorevolmente sul documento è per questo che abbiamo fiducia nell'Italia, nelle imprese e nelle famiglie italiane e, soprattutto, vogliamo determinare le condizioni per generare speranza e futuro nelle giovani

noi voteremo convintamente la risoluzione e ci ritroviamo nel quadro programmatico e nell'analisi proposta dalla NADEF. Vorrei fare alcune considerazioni. Innanzitutto, ci troviamo di fronte ad una robusta crescita, che è andata ben oltre le previsioni del DEF e che ci fornisce un quadro positivo, naturalmente senza trionfalismi e senza sottovalutare i rischi che ancora ci sono. Questo quadro, validato da tutti gli enti e gli osservatori,

sulla strada da intraprendere, sulle scelte fatte in relazione alla gestione della pandemia. Credo che con onestà intellettuale tutti noi oggi possiamo riconoscere che le scelte fatte, prima dal Governo Conte e poi dal Governo Draghi, nella gestione della pandemia si siano rivelate giuste, soprattutto su un punto cruciale: affrontare il problema della messa in sicurezza dal punto di vista sanitario del Paese era la prima e fondamentale azione per la crescita. Così,

delle famiglie e delle imprese è ai livelli massimi degli ultimi anni, anche rispetto agli anni precedenti alla pandemia,

Cari colleghi e colleghe, riconoscerlo senza pregiudizi ideologici è un elemento di valore per tutti noi, per il ruolo delle istituzioni ed anche per il nostro rapporto con i cittadini. Penso, ad esempio, che certe nostre discussioni sul *green pass* siano state superate dalla realtà e dalla volontà dei cittadini di interpretare questa scelta come una chiave fondamentale - vaccino e *green pass* - per la libertà tanto invocata. Fatta questa doverosa e di correttezza rispetto all'analisi di questi mesi, vorrei soffermarmi su due punti. Noi col PNRR, con i tassi bassi di interesse sul debito, con le politiche della BCE, abbiamo un'occasione più unica che rara: avviare il processo di cambiamento e di trasformazione del nostro Paese, ma non dobbiamo sottovalutare i rischi, prima di tutto la pandemia. Avrete letto come me, nel materiale che ci hanno offerto i servizi parlamentari, che nei Paesi poveri il tasso di vaccinazione è al 6 Colleghe e colleghi, nessuno di noi può pensare in modo realistico che gestiamo la pandemia sul piano globale e nei nostri Paesi senza risolvere questo nodo.

dell'Europa insieme agli Stati Uniti, in relazione a *big pharma*, alla produzione di vaccini e alla possibilità di dotare questi Paesi dei vaccini. Attenzione: nessuno si potrà sorprendere, se questo *trend* non si invertisse nei Paesi poveri, del fatto che possa arrivare domani una nuova variante. Il vaccino è decisivo per bloccare le varianti e se non affrontiamo questo tema, non in chiave pauperistica, ma in una chiave vera e strategica di governo della questione, non andremo da nessuna parte. Altro punto centrale la questione del Patto di stabilità e dell'Europa. Comincia proprio in queste settimane - lo ha annunciato il commissario Gentiloni - la discussione sul tema del nuovo patto di stabilità e delle nuove regole. Io credo che l'Italia, come ebbe la capacità di fare il Governo precedente in relazione alle risorse del PNRR, debba svolgere un ruolo decisivo. Credo che abbiamo le carte in regola e abbiamo anche una personalità, il presidente del Consiglio Draghi, che può davvero metterci nelle condizioni di fare un ragionamento non più solo sulle regole, non più solo sul patto di stabilità in quanto tale, ma sulla possibilità, partendo dal PNRR e dalla scelta nuova fatta in Europa, di renderla strutturale e costruire un nuovo percorso. Ad esempio, se la sfida enorme della transizione ecologica rappresenta il futuro delle prossime generazioni e il futuro dell'Europa,

Questo produrrebbe un'innovazione profonda e una sfida per ciascun Paese. L'altro elemento è quello che ci riguarda. Io rimango convinto che, se il PNRR è una grande opportunità, ancora fare uno sforzo per chiarire, prima di tutto, quali sono la nostra strategia e la nostra politica industriale. Da questo punto di vista confesso che vi sono ancora limiti che considero significativi. Oggi - per esempio - discutiamo giustamente di trovare un modo per gestire l'aumento del costo del metano e dell'energia. Ma la via strategica è quella, anche per l'autonomia del nostro Paese in relazione alla grande questione strategica, di fare rapidamente gli investimenti, in chiave di transizione ecologica, nell'ambito delle energie Da questo punto di vista penso che abbiamo bisogno di registrare il dato. Vi sono poi i grandi temi del lavoro e della formazione. non abbiamo bisogno di tornare indietro rispetto a scelte che abbiamo fatto. Io sono convinto che il reddito di cittadinanza sia stato essenziale per reggere una crisi come quella

il grande tema - non chiaro - della spesa corrente. Non vorrei che ritornassimo al periodo antecedente la pandemia. Colleghe e colleghi, se noi investiamo, come abbiamo deciso di fare, di fare, sulla costruzione - per esempio - della rete degli asili nido, dobbiamo sapere che poi dobbiamo trovare le risorse nella spesa corrente per gestire gli asili nido.

investire sulla spesa corrente è un punto strategico. Usciamo dalla logica ragionieristica e costruiamo una strategia.

positivi di crescita che vanno anche oltre le previsioni di qualche mese. Per questo, finalmente sento dentro di me quel pizzico di orgoglio nazionale che vede oggi l'Italia imporsi anche a livello europeo.

è stata la campagna vaccinale. Grazie alla campagna vaccinale abbiamo finalmente un Paese che guarda al prossimo futuro

Tutela della salute e difesa del lavoro devono procedere di pari passo, ma tutto ciò è possibile soltanto se eleviamo al massimo dei livelli la sicurezza sanitaria del nostro Paese. Quindi, oggi rivendichiamo con coerenza di aver scelto questa linea senza alcun ripensamento, e i dati economici ci danno assolutamente ragione. Due giorni fa il Governatore della Banca d'Italia, e quindi non certo un partito politico, ha certificato la crescita del prodotto interno lordo di quest'anno a un fatidico 6

dovute all'efficacia della campagna vaccinale, a cui questo Governo e soprattutto la nostra linea politica hanno impresso un cambio di passo rispetto al passato. Questo è importante. È una premessa che ci tenevo a fare e ad evidenziare. Adesso consideriamo qualche dato, come hanno fatto anche altri colleghi: la crescita del PIL

e imprese. Tornano a espandersi le attività produttive nei settori privati. È chiaro che c'è una forte crescita del settore delle costruzioni e migliorano anche le stime dei consumi privati, al 5,2 "fiducia" sia la parola fondamentale: gli italiani oggi tornano a consumare e a investire perché stanno ritrovando la fiducia nel loro Paese. È questa oggi - secondo me - la marcia in più. Ecco perché dobbiamo continuare a trasmettere

Ci darà una mano sugli investimenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza; ne abbiamo parlato tutti ed è importante per i prossimi anni riuscire a spendere tutte le risorse. Gli investimenti

al presidente Berlusconi, con il Governo di qualche anno fa, che abbiamo abolito l'IMU nel nostro Paese. *(Applausi)*. La casa è la sicurezza primaria degli italiani ed è frutto di una vita di sacrifici.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, sottosegretario Guerra, annuncio fin da subito che il Gruppo Lega voterà

e finanza, che dimostra che l'operato del Governo, delle forze di maggioranza e della Lega all'interno della coalizione di Governo porta a risultati sicuramente migliorativi per l'economia del nostro Paese e crea delle opportunità anche per il futuro. È evidente un dato su tutti: ad aprile prevedevamo nel Documento di economia e finanza una crescita cento, mentre oggi registriamo una previsione finale del 2021 al 6 per cento. Questa è la dimostrazione che le politiche economiche del Governo funzionano e che la lotta alla pandemia

di tutti coloro che si stanno rimboccando le maniche per ripartire a produrre, a lavorare, a creare ricchezza per il Paese. Credo che risultato principale di questo 6 per cento sia legato non strettamente alle politiche del Governo, ma al merito di tutti quei lavoratori, di tutti quei titolari di attività che hanno patito le le chiusure nell'anno passato e che oggi hanno voglia - e lo stanno dimostrando con i fatti, con il loro impegno quotidiano - di risollevare le sorti del Paese. Per noi significa anche *stop* - ci auguriamo sia definitivo - ai decreti-legge sostegni e ristori, che erano evidentemente necessari, ma che hanno rappresentato una spesa considerevole per le casse dello Stato. Quindi, sì al lavoro, sì alla ripartenza, basta chiusura, basta spesa a debito. a debito. Un altro dato importante che fa rilanciare la nostra economia è senza dubbio quello dei tassi di interesse sul debito pubblico che, per quanto cresciuto nell'anno e mezzo passato di 180 miliardi, registra quantomeno un tasso di interesse basso, che ci permette quindi di contenere la spesa del debito complessivo, che rimane - ahimè - pur tuttavia, sulle spalle di tutti gli italiani. Vediamo anche positivamente - è indubbio che ci sia - una crescita di fiducia delle imprese e delle famiglie:

troppo complesse nel nostro Paese. Quindi, la sfida non è vinta, è davanti a noi. Questi investimenti sono necessari, sono una grande opportunità, ma dobbiamo lavorare perché diventino opere pubbliche, lavoro effettivo per le nostre imprese e opportunità per il nostro Paese. Paese. Ci sono altri aspetti positivi che riscontriamo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza: mi riferisco ad alcuni collegati. Mi stupisco che ancora oggi, nel 2021, ci sia chi gridi allo scandalo rispetto alla presenza di un collegato che si riferisce all'attuazione dell'autonomia differenziata, e non solo perché questo tema ha fatto parte di altri Documenti di economia e finanza di Governi passati, ma soprattutto perché c'è ancora un equivoco su quella che è l'autonomia differenziata. Abbiamo sentito i luoghi comuni di sempre; la lotta dell'egoismo dei ricchi contro i poveri: è una sciocchezza. L'autonomia differenziata può appartenere alle Regioni del Nord come alle Regioni del Sud. *(Applausi)*. È un'opportunità che si può cogliere alla quale si può anche non aderire. A me risulta che ci siano Regioni del Nord e del Sud che vogliono intraprendere questo percorso. Un'altra caratteristica dell'autonomia differenziata è che non c'è una sottrazione di risorse da Regione a Regione. L'autonomia differenziata non è una lotta tra Nord e Sud, ma è una richiesta da parte dei territori - potenzialmente tutti - di gestire certi poteri e le risorse che lo Stato già oggi utilizza a livello centrale per erogare quei servizi, trasferendoli alle Regioni. Non c'è sottrazione di risorse nei confronti di un territorio nei confronti di altri, ma si tratta semplicemente della gestione diretta di quelle risorse che oggi gestisce lo Stato a livello centrale con il trasferimento alle Regioni, con le relative competenze. Questo significa libertà e soprattutto responsabilità nella gestione delle risorse. È una sfida in cui noi crediamo. Alcuni territori hanno avviato questo percorso ed è giusto rispettare il voto popolare che in alcuni di essi è stato espresso a stragrande maggioranza, perché è una pietra miliare di democrazia che va rispettata. Mi riferisco in particolare a chi ha voluto dare forza a questo progetto consultando gli elettori che trasversalmente, da destra a sinistra, vi hanno aderito. Questi sono Questi sono i lati positivi, come anche la delega - ad esempio - per una legge quadro sulla disabilità, a testimoniare anche qui l'impegno della Lega all'interno del Governo

e migliorati. Mi riferisco - ad esempio - al reddito di cittadinanza. Partiamo dal presupposto che non si voglia cancellarlo. Va bene, ma va evidentemente corretto perché, così come è strutturato, ha evidenziato dei problemi. I problemi vanno risolti. Non bisogna essere ideologicamente ciechi di fronte ai problemi che ha creato, né di fronte al fatto che in alcuni territori - come credo un po' in tutta Italia - ci sia stata, soprattutto nel momento della necessità della ripresa, in estate, mancanza di manodopera soprattutto nel settore turistico.

giallo-verde. Questo era il primo obiettivo e dovrà essere utilizzato in via residuale esclusivamente per coloro che effettivamente non avevano possibilità di accedere al mondo del lavoro. Deve ritornare ad essere questo o deve o deve diventarlo perché, così come è, non assolve a tale funzione. Per quanto riguarda il tema dei *bonus* in edilizia, è evidente che essi non possono durare all'infinito, ma al tempo stesso

I tempi sono stretti perché in Italia le procedure sono lunghe e farraginose. Tali *bonus* devono quindi rappresentare un'opportunità almeno per qualche anno per sviluppare tutte le potenzialità che possono far scaturire.

della carenza di materie prime, dei prezzi dell'energia e del fatto che stiamo assistendo un ulteriore cambiamento a livello globale in cui l'Asia si accaparra le materie prime, l'energia che serve al proprio sistema produttivo e l'Europa, l'Italia e l'Occidente in generale rischiano anche da questo punto di vista di subire una concorrenza ancora più evidenziata da tali accaparramenti. Serve competitività al nostro sistema produttivo. Bisogna dare risposta alla nuova emergenza che non pensavamo si sarebbe verificata che invece sta creando gravi danni. Mi soffermo in

sarà responsabilità di chi oggi prende una tale decisione. Noi questa responsabilità non ce la prenderemo, perché vogliamo essere coerenti in ciò che crediamo e in ciò che rappresentiamo. *(Applausi)*.

Intendo subito entrare nel merito, perché le difficoltà e le sofferenze indotte al Paese dalla pandemia meritano estrema lucidità di analisi. Ritengo che il passaggio fondamentale della NADEF sia quello in cui il Ministro dell'economia dice testualmente: «Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le politiche invariate e il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, tra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le PMI, all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull'alleggerimento del carico fiscale». *(Brusìo. Richiami del Presidente)*. Che lo si voglia ammettere o meno, parlare di spazi fiscali che permetteranno di rinnovare misure in tema di sanità, efficientamento energetico degli edifici, investimento e innovazione nel Fondo di garanzia per le PMI, significa che il Governo ha capito quanto siano state importanti le misure approvate dal Governo Conte II, con il supporto del MoVimento 5 Stelle, in questi settori. Non dovrebbe essere necessaria una traduzione, ma a scanso di equivoci faccio notare che, in primo luogo, il richiamo al rinnovo di misure in campo sanitario non fa altro che evocare l'ingente incremento di risorse che, durante i Governi Conte, grazie al Movimento 5 Stelle, sono state destinate alla sanità, dopo il precedente decennio in cui lo stesso Servizio sanitario - come hanno mostrato diverse autorevoli ricerche - è stato definanziato per circa 40 miliardi di euro, soprattutto a causa delle scelte distruttive compiute negli anni dell'allora Governo Renzi. il riferimento alla conferma di misure in relazione al Fondo di garanzia per le PMI non fa altro che richiamare il potenziamento di questo Fondo operato dal Governo Conte II, a partire proprio da marzo 2020. alla mano, ad oggi il Fondo ha garantito liquidità al sistema produttivo per oltre 200 miliardi di euro, offrendo una rete di protezione, ma anche di rilancio, indispensabile per far trovare le aziende pronte a sfruttare la ripresa. non siamo in piazza! C'è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto su un argomento importante. C'è un brusìo insopportabile.

misura ideata e introdotta nel sistema economico dal MoVimento 5 Stelle, per spingere l'edilizia virtuosa, la rigenerazione urbana e il risparmio energetico. Anche in questo caso ci soccorrono i dati inequivocabili forniti dall'Enea: da inizio anno i lavori di edilizia con il superbonus ammessi in detrazione hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro, con un incremento del 3.600 per cento dall'inizio. I cantieri avviati sono arrivati a quota 46.000, con un incremento del 2.700 e, dai dati osservati dall'Osservatorio sul precariato dell'INPS, emerge che tra giugno 2020 e giugno 2021, grazie al superbonus, il settore delle costruzioni ha registrato un aumento di 92.000 posti di lavoro, di cui 52.000 a tempo indeterminato. Mi fermo qui, anche se potrei continuare, giusto per sottolineare come sia opportuna e direi dovuta la decisione da parte del Governo di prorogare il superbonus del 110 per cento. Richiamare inoltre - come fa sempre la NADEF - la conferma di misure relative agli investimenti innovativi evoca chiaramente due misure fortemente targate Movimento 5 Stelle, la prima delle quali è il Piano transizione 4.0, uno dei progetti più massicci di sostegno agli investimenti delle imprese in beni strumentali, innovazione e formazione. La seconda è rappresentata dalla costituzione del Fondo nazionale innovazione, che poi ha dato vita al Fondo sviluppo e *startup*, che ha determinato un *boom* di nuove aziende. Come ha certificato "Il Sole 24 Ore" il 10 settembre, nei primi otto mesi del 2021 in Italia sono nate 3.000 *startup,* con un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020.

ci sono altri passaggi che testimoniano quanto sia importante e valida l'eredità del Governo Conte II. A tal proposito, il documento dice testualmente che l'intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Quest'obiettivo è reso possibile da previsioni economiche nettamente migliori del previsto. Un PIL 2021 al 6 per cento rispetto al precedentemente indicato 4,5 è, sì, frutto di un rimbalzo dovuto alla pesante caduta del PIL 2020, ma anche di tutte le misure di protezione e rilancio messe in campo dal Governo Conte II a partire dal marzo 2020. i decreti cura Italia, rilancio, agosto e ristori e la legge bilancio 2021, il Governo Conte II ha messo in campo 110 miliardi di euro a beneficio del tessuto sociale ed economico, a cui si aggiungono i 32 miliardi che lo stesso Governo aveva già approvato per finanziare il primo decreto sostegni, poi approvato dall'attuale Governo.

Colleghi, la NADEF, letta con onestà intellettuale, contiene passaggi inequivocabili che certificano quanto il Governo Conte II sia stato in grado di far trovare il Paese preparato per la ripresa. E questo è un fatto, con buona pace di chi, negli ultimi difficilissimi diciannove mesi, non ha trovato niente di meglio da fare che chiedere, nell'arco di una manciata di giorni, aperture e poi chiusure di esercizi commerciali; passare da sì *green pass* a no *green pass* e far cadere un Governo perché non chiedeva l'attivazione del MES, salvo poi accantonare per sempre lo stesso MES dimostrando, se per caso ce ne fosse stato ancora bisogno, che quell'argomento non corrispondeva a una vera convinzione, ma era solo uno strumento brandito per bieche speculazioni politiche. *(Applausi)*. Il nostro MES è lei, presidente Draghi: questo diceva un esponente di Italia non rendendosi nemmeno conto dell'irridente espressione nei confronti dell'attuale Presidente del Consiglio. Il MoVimento 5 Stelle ha cominciato un percorso di cambiamento. Abbiamo sicuramente fatto errori, ma non abbiamo mai smesso di credere alla possibilità di dare una visione al Paese, per l'Italia e per l'Europa. Sostenendo il Governo Conte, siamo riusciti tutti insieme a ottenere dall'Unione europea il Next generation EU, per la prima volta finanziato da un massiccio piano di emissione di debito comune europeo che per noi vale 204 miliardi di euro da qui al 2026.

Da lì la capacità del Governo Conte II di convincere i *partner* frugali e più riottosi e il successivo decollo del Next generation EU. Il MoVimento 5 Stelle vuole continuare a fornire soluzioni innovative, come quelle puntualmente confermate nella NADEF. In conclusione, voglio ricordare un'altra proposta che da tempo abbiamo messo sul tavolo. Visto l'enorme successo del *super bonus* 110 per cento, che poggia sul principio della cedibilità dei relativi crediti d'imposta, da tempo stiamo proponendo l'estensione di questo principio anche ai crediti d'imposta per gli investimenti delle imprese in Transizione 4.0, piano anch'esso apprezzato dalla NADEF e dall'attuale Governo.

che il Piano di investimenti Transizione 4.0 per le imprese sia fondamentale (al punto da meritare un preciso riferimento all'interno dello stesso documento); se crediamo - come ha fatto l'attuale Governo - che le due misure siano così importanti da meritare un riferimento nel PNRR, allora dobbiamo procedere subito all'estensione in legge di bilancio del meccanismo della cedibilità dei crediti d'imposta Transizione 4.0. Sarebbe una misura in grado di generare ingenti liquidità a beneficio delle imprese, una sorta di superbonus imprese evocato da tutte le principali associazioni imprenditoriali. Non deve essere un dubbio interpretativo di Eurostat o Istat a bloccare una proposta d'investimento che potrebbe mettere l'Italia su quel sentiero di crescita duratura che l'attuale Governo si è dato come obiettivo nella NADEF. Sempre in tema di proposte - per concludere - oggi in audizione il ministro Franco ci ha piacevolmente sorpreso, confermando che il *cashback* ha prodotto effetti positivi e si è rivelato una misura importante per muovere verso i pagamenti elettronici. Ricordiamo che mesi fa anche il Forum Ambrosetti aveva usato parole lusinghiere, pubblicando un rapporto secondo il quale il *cashback* genererebbe oltre 9 miliardi e mezzo di euro di benefici fino al 2025, in termini di riduzione di dell'IVA, di maggior gettito e di emersione del sommerso. Eppure, lo stesso ministro Franco a giugno aveva avallato la sospensione della misura. Riteniamo quindi che il Governo e segnatamente il MEF debbano chiarirsi tempestivamente le idee e recuperare con le opportune correzioni il *cashback*, una misura economica estremamente innovativa ereditata dal Conte II, in grado di sprigionare un elevato potenziale anche per quanto riguarda la digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione. È con questi due ultimi auspici e con la consapevolezza che quanto presenta il NADEF oggi è il frutto di un impegno dei precedenti Governi, che a questo punto non possiamo che ringraziare per l'impegno profuso, che dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

colleghi oltre me, si prefigge di espungere e di stralciare dalla NADEF l'autonomia differenziata. di tale materia in quest'Aula oggi abbiamo parlato in quattro o cinque: noi che abbiamo firmato questo emendamento e la Lega. Detta constatazione dovrebbe essere di per sé chiarificatrice. Tutti gli altri hanno parlato di numerelli; tutti gli altri hanno parlato di altri aspetti importantissimi, ma nessuno ha fatto cenno al fatto che l'autonomia differenziata, che tanti qui dentro hanno avversato giustamente - non ci sono le condizioni non ci sono le condizioni - viene surrettiziamente infilata all'interno del provvedimento in esame. In conseguenza del collegamento con la manovra di bilancio, sarà difficilissimo per il Parlamento e per ciascuno dei parlamentari emendare questo disegno di legge. Non solo: qualcheduno potrebbe anche ritenere che, essendo collegata a una manovra di bilancio, sia materia sottratta anche al *referendum*. Questa è la democrazia diretta dei 5 Stelle. In questo modo voi date onore a quello che avete sempre decantato fino a adesso. Complimenti! Bravi! L'autonomia differenziata, difendete il Sud, "nessuno rimanga indietro": è stato detto dalla Lega nei vari interventi che però non c'è bisogno, perché si compete tutti ad armi pari, partendo a 95 metri su 100. Questa è la differenza.

vi credo più. Se davvero l'avete dichiarato - la vostra faccia dovrà pur rendere conto a voi stessi e al Paese, prima o poi votate per questo emendamento. *(Commenti)*. Mi rivolgo a chi voglio, mi rivolgo all'Aula. Votate questo emendamento, perché si abbia nel Paese una discussione su questa materia. materia. Non è possibile chiuderla in un cassetto e farla approvare di nascosto. Questo state facendo: la state approvando di nascosto. Questo state facendo. E allora *cuique suum tribuere*, a ciascuno il suo: verrà il giudizio del popolo e dovrete rispondere di questo. Dovrete rispondere di una tale nefandezza. "Nessuno rimanga indietro", dicevate. Ecco, voi volete competere ad armi impari con tutti quanti. Bene: votate l'emendamento, stralciate oggi questo disegno di legge dal collegamento con la manovra di bilancio, perché sia poi fatta una norma specifica *ad hoc*, un disegno di legge che fissi ad esempio i

Grazie

Prima di passare agli auspicati interventi di fine seduta, chiedo al Senato

di Eugenio Duca, scomparso improvvisamente ieri mattina. Eugenio Duca è stato parlamentare, deputato della Repubblica dal 1994 al 2006, in un decennio cruciale per la nostra Repubblica. Fu eletto con i progressisti e poi con L'Ulivo, di cui fu uno dei fondatori. Eugenio è stato soprattutto, per tutta la vita, un militante appassionato del movimento dei lavoratori. Ha cominciato le sue battaglie per il lavoro da lavoratore nelle ferrovie e poi da dirigente sindacale nel settore dei trasporti. Ha cominciato da giovanissimo le sue battaglie per i portuali di Ancona e per il porto di Ancona. È stato la voce dell'anima popolare Il suo legame con Ancona è sempre stato indissolubile. È stato abitante di Torrette, un antico borgo di pescatori, stravolto dalle vicissitudini del Novecento, emblema di contraddizioni e trasformazioni; un quartiere cerniera tra la città, la via la via Flaminia e la raffineria di Falconara, un quartiere colpito dalla frana del 1982 e pieno di contraddizioni e di bisogni che Eugenio Duca seppe rappresentare, perché seppe rappresentare le fasce sociali che rischiavano di pagare per un modello predatorio e sbagliato di crescita urbana. Voglio qui ricordare le sue battaglie contro la speculazione edilizia. Tutto questo lo rese amato in città e lo portò in Parlamento. Fu sempre un tenace e inquieto militante della Sinistra; fu sempre molto rispettato nel mondo dei trasporti e della portualità per la sua competenza. Signor Presidente, in queste ore moltissimi sono i cittadini che gli stanno tributando omaggio

Non è questa la politica che vogliono i cittadini e che noi tutti vogliamo. La politica deve essere confronto sui temi, che può essere anche acceso, ma non può essere segnato da atti di violenza, sia fisica che verbale, indipendentemente da chi e a quale forza politica appartenga. Gli attacchi a candidati e a portavoce del MoVimento 5 Stelle rappresentano un segnale pericoloso di un preoccupante decadimento dell'agone politico e la spia di un clima pesante, quasi di odio e di intolleranza, che pervade spesso le consultazioni elettorali. Ciò che è accaduto a Nardò, ad Afragola, a Piedimonte Matese, a Monteparano, a Battipaglia - e l'elenco è lungo è molto grave e pericoloso. Ogni forza politica dovrebbe condannarlo in maniera netta *(Applausi)* e inequivocabile, senza se e senza ma. Piena solidarietà va alle vittime di questi episodi - ribadisco - gravi ed esecrabili. La vera democrazia si fonda sul rispetto delle idee e dei diritti altrui. Attendiamo con fiducia che le Forze dell'ordine completino le indagini e facciano chiarezza sui fatti accaduti. In particolare, alla deputata del MoVimento 5 Stelle di Afragola, Iolanda Di Stasio, che conosco personalmente, ho inviato a nome mio e e di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle del Senato un messaggio sentito di vicinanza e di stima, esprimendole il sostegno e la certezza che quanto avvenuto sarà uno stimolo ulteriore per accrescere la sua forte determinazione e la convinzione di continuare sulla strada intrapresa. Viva la vera politica; abbasso la violenza. Signor Presidente, parto dall'applauso che lei ha sollecitato poco fa. È con grande gioia che ieri mattina ho accolto la bellissima notizia del premio Nobel per la fisica a Giorgio Parisi per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazione nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Giorgio Parisi ha scoperto schemi nascosti in materiali complessi disordinati. Le sue scoperte sono tra i contributi più importanti alla teoria dei sistemi complessi. Esse permettono di comprendere e descrivere molti materiali e fenomeni diversi e apparentemente del tutto casuali, non solo in fisica, ma anche in altri ambiti molto diversi, come la matematica, l'informatica, l'intelligenza artificiale, la mineralogia, la biologia, le neuroscienze e la climatologia. Oltre che essere un importantissimo traguardo personale, rappresenta anche uno straordinario risultato per l'università italiana, per la ricerca nazionale e per l'intero sistema Paese.

Le geoscienze sono nella nostra quotidianità e rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile, a livello economico, sociale e ambientale, del nostro Paese; riguardano risorse idriche, minerarie, energie, dinamica fluviale e costiera, protezione dai rischi geologici e idrogeologici, sicurezza ambientale e salute umana. La settimana del pianeta Terra vuole far conoscere al grande pubblico le geoscienze, attraverso lo straordinario patrimonio geologico, ambientale, naturalistico e culturale del nostro Paese, toccando anche temi diversi: cura e salvaguardia del territorio, tutela dell'ambiente, mutamenti climatici in atto, sviluppo ecosostenibile, transizione ecologica, rischi connessi ai pericoli naturali, turismo culturale sensibile ai valori ambientali. Con questo obiettivo, dal 3 al 10 ottobre 2021, nell'ambito della nona edizione della Settimana del pianeta Terra, si svolgono in Italia tanti tanti geo-eventi: escursioni, passeggiate nei centri urbani, porte aperte nei musei, centri di ricerca, osservatori astronomici, laboratori didattici e sperimentali, esposizioni e mostre; convegni, attività artistiche e musicali. Contiamo di avvicinare qualche futuro Giorgio Parisi.

- come noto - non si è mai risparmiato, soprattutto negli ultimi due anni, per garantire gli approvvigionamenti di cibo e soprattutto di prodotti di qualità. La filiera lattiero-casearia italiana vale 16 miliardi di euro di giro d'affari, con oltre 100.000 addetti al settore. Esiste un notevole divario, però, in questa filiera tra i prezzi all'origine e quelli al consumo. Per quanto riguarda il mercato del latte *spot*, ad esempio, la quotazione è di circa 41 centesimi; quello sotto contratto, vale a dire quello ritirato quotidianamente dai caseifici per la produzione di latte fresco e formaggio, vale dai 35 ai 37 centesimi I bilanci 2020 della grande distribuzione organizzata evidenziano un forte recupero di marginalità rispetto all'anno precedente. Gli allevatori, che sono l'anello debole della filiera, avendo uno scarso potere contrattuale, vedono sempre più ridursi i loro profitti; anzi, in molti casi, i costi superano i ricavi. Gli allevamenti sono inoltre sotto pressione a causa dell'aumento dei prezzi dell'alimentazione, dei foraggi, del mais, della soia, e soprattutto per l'aumento dell'energia elettrica, delle materie prime, della logistica e dei trasporti. Nei contratti di fornitura tra la grande distribuzione organizzata, le industrie di trasformazione e gli allevatori devono essere concordati compensi equi, che possano assicurare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti, sottraendoli al rischio del fallimento. È assurdo e vergognoso che tre litri di latte valgano quanto una tazzina di caffè. Questo è inaudito. Il mancato accordo, poi, proprio in questi giorni, sulla firma del protocollo d'intesa al Ministero delle politiche agricole, che coinvolge tutta la filiera del latte, non apre a segnali incoraggianti per il futuro, lasciando il settore in preda a uno stato di sofferenza che va ad alimentare una crisi più ampia e strutturale, in cui stanno affondando i nostri allevatori e produttori di latte. Da quest'Aula il nostro è un grido e un appello forte e immediato, affinché il Ministro delle politiche agricole non attenda ulteriormente, convochi immediatamente il tavolo di filiera e trovi una soluzione adeguata, affinché ogni componente della filiera possa vedere equamente redistribuito il ricavo e, di conseguenza, la marginalità, che per le stalle italiane rappresenterebbe semplicemente l'ancora di sopravvivenza. *(Applausi)*.

ha causato un'alluvione importante, anzi importantissima, che ha toccato e messo in ginocchio molti Comuni e soprattutto tutta la macchina della Protezione civile, che non si è fermata un secondo. A volte queste previsioni non sono così facili da fare e la forza della natura ci ha dimostrato ancora

si è dato un gran da fare. Purtroppo però a volte capita che ci siano degli incidenti e quest'uomo è rimasto sotto l'acqua dell'alluvione con il trattore ribaltato e ha rischiato di perdere la vita. Vorrei allora fare una riflessione, signor Presidente, non solo rispetto a queste occasioni, ma in generale sui sindaci, che tutte le volte sono in prima linea, tutte le volte dimostrato grande capacità di

dicendo che aziende importanti sono state messe in ginocchio, soprattutto nella zona del confine tra il Piemonte e la Liguria; nell'ovadese in un'azienda faunistica venatoria sono morti nell'alluvione circa 5.000 capi. Questo è inaudito e credo che su questo il il Governo dovrà porre attenzione nel momento in cui la Regione chiederà lo stato di calamità.